con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Senatori, desidero rivolgere un pensiero di commossa partecipazione al dolore dei familiari, dei colleghi e degli amici del senatore Luigi Covatta. Giornalista, scrittore, politico, uomo delle Istituzioni, Luigi Covatta è stato una delle voci più autorevoli del socialismo italiano, un riformista per indole e vocazione culturale. Acuto osservatore delle dinamiche sociali ed economiche del Paese, fu tra i primi, nel finire degli anni Sessanta, a suggerire l'idea di un contenitore politico che potesse riunire e rappresentare i cattolici progressisti di sinistra: un'idea che Luigi Covatta sostenne con ferma convinzione, prima nella breve avventura del movimento politico dei lavoratori, e quindi nell'instancabile impegno anche culturale all'interno del partito socialista italiano, italiano, di cui è stato per quasi vent'anni uno dei principali esponenti dell'ala più riformista e riformatrice. La stessa attenzione con cui, Eletto per la prima volta alla Camera dei deputati nel 1979, Luigi Covatta è stato parlamentare per ben quattro legislature, di cui tre qui in Senato, e più volte Sottosegretario di Stato sia alla pubblica istruzione che ai beni culturali e ambientali, incarichi ricoperti sempre con rigore, responsabilità, fermo rispetto per le istituzioni e soprattutto grande attenzione alle istanze dei cittadini e della società. La stessa attenzione con cui, anche dopo essersi ritirato dalla politica attiva ed essere tornato all'editoria, Luigi Covatta ha continuato a osservare, interpretare, spiegare e raccontare tante pagine della nostra epoca, sempre con intelligenza, acume, ironia, libertà e onestà di pensiero, doti per le quali nel 2009 era stato chiamato a dirigere «Mondoperaio», storica rivista socialista fondata da Pietro Nenni, che Luigi Covatta ha contribuito a rilanciare, consolidandone il prestigio come autorevole incubatore di idee e di iniziative culturali. È di questi giorni la notizia che la biblioteca del Senato sta ultimando i lavori di digitalizzazione, iniziati lo scorso anno, dell'intera collezione della rivista sin dal primo numero, un progetto a cui lo stesso Luigi Covatta aveva aderito con entusiasmo e attiva partecipazione. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata motivo di profondo dolore per tutti, perché ci lascia orfani di una personalità forte e di grandi valori. Un intellettuale di carisma, sensibile e generoso, sempre schierato al fianco dei lavoratori; un politico appassionato, con una fede incrollabile nelle proprie idee, ma sempre pronto al confronto e alla dialettica costruttiva, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle ragioni di tutti. In ricordo del senatore Luigi Covatta invito pertanto l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

per alcuni potrebbe sembrare sorprendente l'eco suscitata in questi giorni dalla scomparsa di Gigi Covatta: i messaggi di cordoglio pubblici, gli editoriali di ricordo e di riflessione, il sentimento che ha attraversato vecchi e giovani compagni socialisti, ma anche personalità distanti dalla sua formazione, sono ben lungi da ciò che tradizionalmente si riserva a un ex parlamentare. La verità è contenuta nei suoi scritti, da lei ricordati, sulla rivista «Mondoperaio», nella qualità e nell'attualità dei suoi ragionamenti, nella penna fine e preziosa con cui li scriveva. La verità è questa: Covatta fu un politico e un intellettuale antico nella militanza totalizzante, fatta di confronti infiniti, di sigarette mai spente, di passioni mai sopite, di aneliti mai domi, e fu moderno nella capacità di lettura dei fenomeni, nell'intuizione riformatrice, nella contaminazione ardita. Fu anomalo nel suo essere cristiano e socialista, quando i cristiani avevano una casa ineludibile e i socialisti sapevano di laicismo sferzante. Una vita di feconde contraddizioni, quella di Covatta. Fu militante nell'Associazione cattolica contro il doroteismo democristiano; fu socialista lombardiano, ma criticamente al fianco e mai contro la modernizzazione di Bettino Craxi e fu uno degli ispiratori del Manifesto di Rimini i meriti e i bisogni. La sua levatura fece il paio con un tratto umano di una sincerità disarmante che solo un intellettuale vero e onesto sa avere. polemista, ma mai polemico; sapeva negare nell'ironia i suoi disaccordi e nella parola scritta trovava il grimaldello ideale per scardinare totem e tabù. Insomma, diciamocela tutta, non c'entra nulla con l'attuale tempo politico, fatto di leggerezze al limite dell'inconsistenza, di forme senza sostanza, di decisioni senza pensiero. È per questo, forse, che lo ricordiamo tutti oggi con ammirazione e sentimento, ai quali personalmente affianco l'amicizia e la consonanza di compagno di mille battaglie, di mille condivisioni, anche di qualche discordia, quando la politica aveva la "P" maiuscola e cambiare la società impegnava tutta la vita. Ciao Luigi!

Signor Presidente, ho conosciuto Luigi Covatta quando nacque l'Ulivo e lui fu attivissimo, ma discretissimo. Gli interessavano i contenuti e i programmi, non le foto con i protagonisti di quella stagione. L'interesse per l'importanza dei contenuti della riforma lo testimoniava anche adesso con il suo impegno per una riforma costituzionale per, come aveva detto lui, cicatrizzare il taglio dei parlamentari, per correggere e non demonizzare una riforma.

sempre motivato, competente e un lavoratore instancabile, mai domo, anche quando la politica gli ha riservato profonde delusioni, come nelle elezioni del 1972 e, via via, lungo tutto il suo percorso nel Partito Socialista Italiano, come è appena stato ricordato. Nella sua attività parlamentare e di Governo non è stato mai Ministro, ma sempre protagonista intelligente e determinato, capace di lasciare il segno nelle cose in cui era impegnato. presidente di «Italia Lavoro» e ricordo, inoltre, la sua capacità di scrivere, di spiegare, di razionalizzare. Fece risorgere «Mondoperaio» e ne diventò direttore e mi piace qui riprendere una definizione usata dalle ACLI di Milano per ricordarlo: «Moderatamente rivoluzionario, rivoluzionariamente moderato». Esprimo un saluto commosso e una partecipazione sincera al dolore dei tuoi cari e dei tuoi compagni di strada, carissimo Luigi.

Per trovare Gigi bisognava seguire le tracce del fumo delle Gauloises o, in alternativa ai portaceneri strapieni di Gauloises, infilarsi in una libreria. Gigi viveva tra sigarette fumate a metà, come ricordava prima l'amico Pittella, e libri. Era un autentico oppositore del presentismo ed era soprattutto un intellettuale napoletano raffinato che continuava a convincerti che la politica è un mestiere, ma per essere tale bisogna farla come tutti i professionisti. Bisogna studiare, studiare e studiare, leggere, leggere e leggere, approfondire, approfondire cosa che oggi forse non è più considerata assolutamente adeguata. Ha avuto una storia piena; con lui demmo vita alla seconda fase di «Mondoperaio» nel 2009, come lei ha ricordato. Ma anche la sua storia precedente è decisamente interessante. Apparteneva a quell'anima cattolica-sociale, che arrivò al PSI all'inizio degli anni Settanta; arrivarono in molti, ma soprattutto lui, Livio Labor e Gennaro Acquaviva. Vi arrivarono perché avevano individuato nel socialismo umanitario la possibilità di coniugarvi, nella maniera politicamente più perfetta possibile, la dottrina sociale della Chiesa. Da allora non hanno mai abbandonato questo destino, ma l'hanno coltivato con serenità. Era il tempo in cui i fermenti nel mondo cattolico erano una sorta di tempesta quotidiana; era il tempo in cui Gigi Covatta parlava a lungo, con quella esperienza della Barbiana che aveva avuto alla testa don Milani. Era un uomo di minoranza, come tutti gli intellettuali, anzi se ne vantava. Il libro in cui confidava di più aveva espressa già nel titolo la sua appartenenza: era «Menscevichi»; e i menscevichi, come noto, sono la minoranza rispetto ai bolscevichi, Quei menscevichi erano i riformisti nella storia dell'Italia repubblicana e prerepubblicana, sempre, costantemente in minoranza, da cattolico eretico - perché fece una scelta fuori dalla Democrazia Cristiana - e in quanto appartenente a una storia, quella socialista, che dal dopoguerra, nella sinistra italiana, aveva rivestito e occupava quella dimensione. Se, però, Gigi ebbe un ruolo (e lo ebbe un ruolo (e lo ebbe veramente), fu quello (e fu uno dei pochi) di fornire munizioni all'allora segretario Bettino Craxi (e furono munizioni pregiate) per contendere al Partito Comunista Italiano l'egemonia culturale nella sinistra. Chi ha giudicato quella storia, in maniera diabolica, come storia di nani e ballerine ha dimenticato che il mondo che Gigi Covatta mise in movimento attraverso la prima fase di «Mondoperaio» aveva nomi che hanno fatto la storia della cultura italiana: erano Amato, Vassalli, Massimo Severo Giannini, Cheli, Cassese, Reviglio, Lina Wertmüller, Mario Soldati e, poi, Gassman, Gianni Brera, Federico Zeri e moltissimi altri. Altro che nani e ballerine! Era una storia che si rivelò, alla fine, a suo modo vincente, perché impose nella sinistra italiana, grazie a Gigi, una visione riformista che non le era assolutamente propria. propria. Ricordo volentieri che la seconda vita di «Mondoperaio», che lui guidò, la affidò soprattutto a un mondo che è presente anche qui in Aula, una nuova generazione, e lo fece sulla base della coerenza. Ecco, trovo ancora che la coerenza sia un valore. Quella di Gigi fu una coerenza condotta fino alla fine dei suoi giorni.

Con Covatta scompare un importante dirigente del Partito Socialista Italiano, un grande intellettuale, un riformista autentico, protagonista della vita politica. ha già detto chi mi ha preceduto, a noi spesso capita di ricordare personalità politiche. Forse da questo punto di vista potremmo dire che una riflessione oggi è doverosa. Lo spessore e la qualità politica di personalità come Covatta ci dovrebbero stimolare a uno sforzo, a un colpo di reni, al di là delle posizioni politiche e culturali, per dare alla politica quello spessore che, soprattutto in un momento come questo, merita ed è, anzi, essenziale per assicurare qualità alla democrazia. In quegli anni fu protagonista in primo luogo con le ACLI, sostenendo con forza l'unità sindacale, il nuovo statuto dei lavoratori. Nel 1969 fondò, con Riccardo Lombardi, un'associazione

le elezioni politiche del 1972, dove il Movimento Politico dei Lavoratori non ebbe un risultato positivo, Covatta, insieme a tanti suoi colleghi, aderì al Partito Socialista. Ne fu capo dell'ufficio studi nel 1979; ha assunto incarichi di Governo, incarichi istituzionali. Il suo protagonismo è certamente importante, come è stato ricordato, con l'obiettivo di mettere in discussione la cosiddetta egemonia culturale del Partito Comunista. Diede un contributo importante al progetto socialista del 1978 e all'Alleanza riformatrice dei meriti e dei bisogni della conferenza di Rimini del che - voglio dirlo - per me rappresenta una delle elaborazioni più interessanti e innovative di quegli anni e uno stimolo a una riflessione che - ahimè - la sinistra nel suo complesso non riuscì a fare. Non voglio negare la dialettica - io ero su posizioni diverse ma certamente riconosco che, da quel punto di vista, fu fatto un lavoro importante. In conclusione, voglio fare una breve riflessione sul concetto di riformismo.

Insisto: siamo in una fase nuova; è cambiato tutto. Ragionare e avere l'ambizione culturale, politica e storica di essere riformisti significa avere il coraggio di una nuova radicalità, un nuovo modello di sviluppo, una nuova idea di società. Questo è il riformismo, perché senza una visione ampia il riformismo rischierebbe di diventare una pratica amministrativa. E pur da posizioni diverse,

non è facile ricordare, senza cadere nella retorica, una personalità scomparsa. Lo è ancor di più se bisogna commemorare un socialista, un intellettuale inquieto ed eretico, dal carattere schivo e introverso, come è sempre stato Luigi Covatta. Ironico e autoironico, Gigi, come era affettuosamente chiamato da amici e compagni, è stato una tessera brillante di un mosaico di intelligenze che contribuì allo sviluppo di quel nuovo corso socialista che ha rappresentato, nonostante una certa lettura faziosa che egli ebbe sempre a contrastare, un fattore fondamentale del progresso italiano. Infatti Covatta dopo un'avventura significativa dal punto di vista culturale, ma assai scarna di risultati, come fu quella del Movimento un movimento cattolico riformista - di fatto una delle esperienze più interessanti della presenza cattolica nella politica militante - aderì con un manipolo di intelligenze dopo le elezioni politiche del 1972 a un Partito socialista in preda ad una profonda crisi culturale, ancor più che strategica ed elettorale. Si trovò così, prima a fianco di Riccardo Lombardi, poi di Bettino Craxi, ad essere quello che io amo definire un intellettuale di campo. Come è proprio di chi ha cultura riformista, si sporcò le mani, sperimentò le difficoltà e le asprezze della politica, non limitandosi a una sola elaborazione teorica, ma svolgendo all'interno del partito e delle Istituzioni un'azione forte, talvolta controcorrente come era uso fare in una casa libertaria qual è quella socialista, fungendo così da raccordo fra il variegato mondo intellettuale che ruotava intorno a Craxi e i socialisti. Covatta è stato inoltre uno dei protagonisti principali di quella ineguagliata Conferenza programmatica di Rimini del 1982, tanto come ideatore che come relatore. A lui infatti fu affidata la relazione introduttiva che schiudeva le porte a una nuova fase socialista con un passaggio - si diceva allora - dal progetto al programma, ponendosi il tema della governabilità del Paese. Governare il cambiamento fu il motto e la missione socialista di quegli anni che, come asseriva Covatta nel suo intervento, non è non è pretestuoso mettere al centro del programma socialista unitamente a quel messaggio riformista che individua nella società i nuovi soggetti dell'innovazione e del progresso politico. Covatta, al pari di molti ragazzi della sua generazione, di ogni colore e parte, ha inteso la politica, quella politica che oggi rievochiamo con l'uso enfatico della "P" maiuscola, come il terreno di gioco cui dedicare la propria vita, un campo di gioco da cui non uscì neanche dopo la distruzione della casa socialista, avvenuta all'interno di quella falsa rivoluzione che prese il nome di "tangentopoli" e dopo la conseguente fine della sua esperienza parlamentare. La sua esperienza e quella di tanti ci deve ricordare che la politica, la buona politica non può e non deve esaurirsi nella pratica parlamentare di cui è solo una parte. Ha così scelto nella seconda Repubblica di cimentarsi in un'opera di lettura e di rilettura dell'epopea craxiana, contribuendo, al pari di tanti altri compagni, a impedire la *damnatio* *memoriae* di una storia di civiltà

Ricordo una cena a Bari, qualche anno fa, in cui dibattemmo fino a tarda sera tra un bicchiere di vino e molto di più di qualche sigaretta, su alcune vicende della nostra storia. Ho riconosciuto in lui lo spirito libero, l'intellettuale autocritico, prima che criptico, e ho sempre condiviso uno dei suoi crucci da Rimini a oggi, passando per la tragica legislatura 1992-1994, quando ricoprì l'incarico di vicepresidente della Commissione per le riforme istituzionali: la necessità di dare vita ad una profonda riforma istituzionale di cui nessuno parla e di cui oggi, ancor più di ieri, abbiamo un disperato bisogno. È un nodo irrisolto che a causa della lunga e perdurante crisi italiana*... commentatore attento e acuto qual era non ha mai fatto mancare la sua voce. Onorevoli colleghi, salutare un compagno, dare l'ultimo commiato a un membro della propria comunità, perché i partiti erano innanzitutto questo, è doloroso, credetemi, ma sono fiduciosa che Gigi continuerà a vivere nella memoria di tanti, nei suoi scritti e nelle sue carte, e che in questo momento, ovunque lui sia, ci starà guardando sornione, fumando la solita sigaretta.

Signor Presidente, non conoscevo il senatore Luigi Covatta se non indirettamente per i suoi scritti, ma anche per le sue origini. Covatta era campano, era nato a Ischia, e leggendo le sue opere si scorge nel suo lavoro, nel suo approccio,

repubblicana». Sappiamo che i menscevichi sono i perdenti della rivoluzione russa, sono i riformisti democratici che perdono la sfida con la storia, sopraffatti dal colpo di Stato di ottobre dei bolscevichi. titolo non casuale, che esprime un'amarezza, la percezione che la Sinistra cattolica italiana riformista e i suoi obiettivi avevano perso la sfida con la storia in un determinato periodo della nostra Italia. È interessante ricordare Covatta facendo riecheggiare in quest'Aula le sue parole di un suo scritto del 2007, 2007, che è ancora legato ad una stagione superata, ma di cui sopravvive lo spirito. Consentitemi di leggerne un breve passo: la partitocrazia in Italia - scrive Covatta - non è calata dal cielo, né si è conformata, come ritiene una discutibile vulgata, principalmente agli orientamenti delle potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale. Lucio Caracciolo - scrive Covatta -, che pure definisce l'Italia postbellica un semiprotettorato, tiene a precisare che un semiprotettorato non è una colonia né un palatinato; per cui, benché condizionata, consociata, la Prima Repubblica è restata comunque e prima di tutto una democrazia, in cui i Governi italiani sono stati scelti dagli italiani e non dagli americani. Questa è una frase sintomatica del pensiero di Covatta, perché ci sta dicendo che noi non siamo vittime della storia; ci ricorda che ne siamo gli artefici. Nello spirito di Covatta c'era la percezione di una tragedia che riguarda il nostro Paese e la nostra politica; la tragedia data da una democrazia bloccata, dove ancora oggi ci portiamo dietro il retaggio, che secondo lui probabilmente trova le radici nell'esperienza fascista, per cui l'avversario è un nemico. Forse è questo il grande insegnamento che Covatta ci lascia ancora oggi, è il motivo per cui le sue opere sono ancora vive anche se scritte in anni ormai lontani, apparentemente lontani. La sua è un'opera ancora viva, perché ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Se lui fosse qui oggi e potesse osservare quanto sta accadendo probabilmente ci direbbe: ricordatevi che oggi, in questo momento più che mai, in un momento di grande cambiamento, anche per un fattore esterno qual è la pandemia, voi avete nelle vostre mani il futuro del Paese, ma per portarlo a essere moderno ci ricorderebbe che dobbiamo riconoscere gli uni negli altri avversari e non nemici. Signor Presidente, ho chiesto a lei questa mattina di intervenire sull'ordine dei lavori, perché la Lega desidera affrontare pubblicamente una situazione politica che è meglio che ci diciamo tutti quanti e che intendo comunicare anche a lei che è la seconda carica dello Stato. È da più di un mese, da quando è nato questo Governo, che chiedo espressamente una riunione con tutti i Capigruppo di maggioranza per decidere quali sono i disegni di legge da calendarizzare nelle varie Commissioni. La risposta, dopo un mese e mezzo, è quella che in ogni singola Commissione la vecchia maggioranza (poi deciderete voi se è legittimo o meno), è legittimo o meno), quindi la maggioranza dell'attuale maggioranza, vuole andare avanti a calendarizzare disegni di legge identitari e in molti casi divisivi.

sotto l'aspetto sanitario ed economico, di accantonare - ha usato questo termine - tutto ciò che ha significato un marcare la differenza tra i vari partiti negli ultimi venti anni.

una mozione che era stata presentata e aveva avuto una votazione differente, pur essendo una mozione, perché ha specificato che in questo momento i cittadini hanno bisogno di fiducia. E la fiducia, come gliela diamo? Essendo tutti uniti sui temi emergenziali di adesso, non solo al Governo, ma anche al Parlamento. Di fronte a queste parole, di cui ho preso anche nota, il risultato allora è quello che vedo: nel Parlamento si va avanti e la vecchia maggioranza va avanti come se al Governo ci fosse ancora Conte. Ripeto: prendo atto di questo, però è anche ora che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità davanti al Governo e davanti al presidente Mattarella che ha voluto questo Governo e ha voluto questo momento. *(Applausi)*. Andare avanti con questi temi divisivi significa avvelenare il clima all'interno e mettere in difficoltà e ulteriormente a rischio una situazione che è già difficile tra di noi, diciamocelo, perché facciamo fatica a trovare l'accordo su tanti temi. Quindi, l'importante è che uno si assuma questa responsabilità. Cosa facciamo, invece? Mentre al Governo si fanno in quattro per sistemare le questioni e trovare l'accordo tra di noi e andare avanti per far uscire il Paese dalle emergenze, noi cosa facciamo in Parlamento? Scateniamo degli incendi nelle varie Commissioni o in Aula su temi che oggi si chiamano Zan, domani sarà lo *ius soli* e poi ce ne saranno altri? No, penso che questo non sia assolutamente possibile, nel rispetto di ogni singola idea. Noi non abbiamo posto il tema dell'affido condiviso, che sappiamo creare problemi, o quello dei decreti sicurezza. Non abbiamo posto altri temi, come la *flat tax*, ma li abbiamo accantonati. Noi abbiamo proposto disegni di legge che non creano problemi a nessuno, che possono essere utili in questo momento di crisi e che possono anche dare - così ce lo diciamo - visibilità e ruolo al Parlamento. Però, scusatemi, la risposta che ci è stata data da parte vostra è davvero negativa sotto questo aspetto. Voi volete portare avanti i vostri temi di bandiera. Ostellari, che poi è stato messo sotto accusa, ha usato solo un po' di responsabilità e buon senso. *(Brusio)*. Scusate, per favore, chiedo di parlare; poi ascolterò quello che dite voi. Il senatore Ostellari ha detto: come maggioranza trovatevi e decidete, perché arrivare ad una calendarizzazione, dove una parte della maggioranza vota a favore, una parte vota contro e si spacca la maggioranza, può creare delle tensioni. È stato attaccato come se Ostellari volesse fermare qualcosa. Nessuno potrà fermare quello che è previsto nel Regolamento. Quindi alzerete la manina e farete quello che dovete fare. L'importante è che ognuno di noi si assuma le proprie responsabilità. *(Applausi)*. Mi avvio Mi avvio alla chiusura: qui il tema divisivo non è l'omotransfobia, su cui siamo tutti d'accordo. Anzi, lo stesso senatore Ostellari si è reso disponibile a modificare l'articolo 61 del codice penale, per aumentare le pene per coloro che discriminano per orientamento sessuale. C'è il tema dei futili e abbietti motivi, ma non solo.

Lo diciamo ad artisti, a presentatori televisivi, a tutto il mondo dei media: la Lega c'è. Cosa è divisivo? Il disegno di legge Zan! Ma non è solo divisivo con noi, ma è divisivo anche a sinistra,

Questo è il tema

Per cortesia, fate terminare. Siamo in un libero Parlamento. ROMEO Il tema del reato di opinione: rispetto le idee LGBT, però voglio che anche gli altri rispettino le mie. Non posso essere messo un domani nelle condizioni di essere bollato, sanzionato, di non potermi candidare, solo perché ho osato contraddire

Ultima questione: il tema della scuola. Nella scuola non voglio che venga imposto un modello, che sia il modello LGBT o che sia il modello Pillon.

divisivo! Oggi si chiama Zan, domani si chiamerà in un altro modo, l'importante è che sia chiaro, davanti al presidente Draghi e al Presidente della Repubblica, chi ha ha appiccato l'incendio in questo Parlamento e in questa fase delicata della nostra Repubblica, senza capire qual è il senso di questo Governo.

Presidente, apprezzo il fatto che il presidente Romeo abbia voluto fare una discussione nella quale ha inserito anche il disegno di legge Zan: noi non stiamo chiedendo altro che fare questa discussione nella sede opportuna, cioè in Commissione.

di cui anche nei mesi scorsi si è tanto parlato. Oggi che c'è un'opportunità in più, vista anche l'ampia maggioranza per poter affrontare i decreti, si tratta di lavorare sui disegni di legge che possono tranquillamente consentire un dibattito nelle sedi opportune. allora al presidente Romeo, senza voler fare una discussione direttamente con lui, che il senso di responsabilità è anche questo, vale a dire che le regole e il Regolamento vengano rispettati. Abbiamo chiesto la calendarizzazione nuovamente, per l'ennesima volta, del disegno di legge Zan: il presidente Ostellari ha deciso di intraprendere un altro percorso che, dal nostro punto di vista,

purtroppo c'è chi lo ostacola in questo modo - è un provvedimento contro i crimini d'odio e io immaginavo che, rispetto alla lotta contro i crimini d'odio, la trasversalità potesse essere completa e totale. *(Applausi)*. Dovremmo infatti imparare anche a chiamare le cose con il loro nome e a non usare solo *slogan* che sono facili nella comunicazione, fermo restando poi che, quando si tocca l'argomento della scuola, bisognerebbe sapere anche come la scuola funziona e sapere che qualsiasi attività viene proposta all'inizio dell'anno, attraverso un patto di corresponsabilità,

è stata sollevata dal presidente Romeo - non è solo il disegno di legge Zan. Il fatto è che tutte le volte che si provano a proporre dei disegni di legge, che magari sono stati già approvati in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento e che quindi qui

deve essere chiaro alla Lega che un Paese, grazie ai sostegni e ai sussidi, sopravvive, ma un Paese cresce se crescono i diritti sociali ed economici dei lavoratori, se si rafforzano i diritti fondamentali della persona. *(Applausi)*. È così che cresce una Nazione. Prendo atto della situazione emergenziale, delle parole del Presidente, ma non c'è Paese al mondo che possa rinunciare a crescere sul tema dei diritti civili della persona, di un individuo.

che una persona possa essere insultata o picchiata semplicemente per il suo modo di essere.

Ostellari, di trovare le giuste declinazioni per interpretare al meglio il sentimento della Nazione. Non sappiamo per quanto tempo ancora dovremo sostenere il reddito di chi il reddito lo ha perso o la liquidità delle imprese che sono in crisi, ma sappiamo che tra un mese le nostre imprese saranno chiamate a sfide straordinarie, dovranno tornare nei mercati esteri e competere con le loro concorrenti, ma per fare questo e per riuscire in questa sfida, hanno necessità di avere alle spalle, da qui al prossimo anno, un Paese finalmente moderno, finalmente moderno, veloce, snello, agile, un Paese che si affacci al millennio della transizione ecologica. Con i suoi discorsi, non andremo da nessuna parte, torneremo solo indietro, torneremo solo indietro, se vogliamo prendere la Polonia come modello di società civile, che bandisce l'identità di genere e che non permette alle persone di frequentare certi luoghi.

senatore Romeo, ieri non ha applicato i principi della democrazia, alzandosi dalla poltrona e lasciando l'ufficio.

Nessuno, nessuno, nessuno può disapplicare il Regolamento del Senato. *(Applausi)*.

Poi sarà l'espressione della volontà dei parlamentari a decidere, ma non lo può decidere né il presidente Ostellari né la Lega: lo deve decidere il Senato, il Senato, soprattutto quando si tratta di temi così importanti.

Abbiamo anche assistito a professioni di ecologismo e di europeismo dell'ultimo minuto pur di entrare nel Governo che dovrà gestire queste risorse.

vediamo i fatti! Noi vi aspettiamo ai fatti! Vediamo se, dietro quelle professioni di europeismo e di ecologismo, ci sono i fatti. Il modo per cui queste verifiche possano essere compiute è solo uno: vedersi qui in Aula e guardarsi in faccia. *(Applausi.

la dignità di tutti i singoli senatori, di ogni forza politica, di ogni Gruppo parlamentare. La libertà del Parlamento, La libertà del Parlamento, che è una libertà anche dai Governi e dalle maggioranze, è quella di esercitare fino in fondo la propria attività legislativa, perché questa è la competenza esclusiva del Parlamento. Se noi mettiamo in discussione questo, mettiamo in discussione l'essenza stessa dei Parlamenti democratici.

nessuno può avere potere di veto. Tutti possono avere, ovviamente, l'obbligo e la facoltà di discutere, di cambiare, di agire per modificare le iniziative legislative e le leggi. Io e larghissima parte dei miei

e della Commissione di inchiesta sulle *fake news*, è dovere di questo ramo del Parlamento esaminarli.

portiamolo direttamente in Aula. Qui nessuno sta mettendo in discussione il fatto che ognuno possa avere opinioni legittimamente diverse

Quello che non è ammissibile è che all'interno di una Commissione dove si registrano pareri diversi il Presidente non porti il disegno

Anzitutto non si può parlare fuori microfono. La parola la do esclusivamente io. Leggete il Regolamento!

Questo è un comportamento di civiltà istituzionale. Prego,

giustamente - pareri e opzioni diversi e quindi si discute nel merito e non attraverso un'attività preventiva ostruzionistica. Questo non è accettabile. Presidente, dovremmo dire che questo passaggio di Governo ha significato che il Parlamento è stato commissariato? Perché questo vorrebbe dire. Penso che nessuno di noi potrà mai accettare che, in una Repubblica libera e democratica, il Parlamento sia commissariato.

io credo che questa mattina stiamo scivolando in una polemica che la natura di questo Governo non merita. *(Applausi)*. Forza Italia non prende lezioni di tutela dei diritti fondamentali da nessuno. E ve lo dice una persona - parlo per un momento a titolo personale - che ha sempre avuto una posizione molto definita e mai nascosta

non accettiamo lezioni di tutela dei diritti fondamentali da chi nella scorsa legislatura ha votato contro le unioni civili e ora si scopre paladino delle libertà. Non accettiamo lezioni di diritti. *(Commenti del senatore Airola)*. Collega Airola, poi faremo un *summit*, lei e io, e ci racconteremo tutto; ma adesso il tema è un po' più alto. Non accettiamo lezioni da chi è entrato a fare parte di una maggioranza che - colleghi, vi do una notizia - non è il Governo Conte; non c'è più il Governo Conte, questo non è il Governo Conte. Non è un Governo politico, è un Governo di unità nazionale, direi di salute pubblica, che mette insieme quello che insieme non starebbe mai, per obiettivi molto definiti: uscire velocemente dalla pandemia, dare ristori a chi ne ha bisogno e fare il *recovery plan*. *(Applausi)*. Lo ripeto: ve lo dice una persona che ha le idee molto chiare sui diritti fondamentali, bisogna rispettare la possibilità di questo Governo di tenersi insieme. Noi non stiamo dicendo che non vogliamo trattare questi temi, ma diciamo che ne vogliamo discutere con voi e che non accettiamo imposizioni. Vogliamo riunioni di maggioranza in cui decidiamo insieme quale sarà il calendario; non possiamo andare avanti a botte di colpi di mano. *(Applausi)*. Tutti gli altri temi, quelli importanti, quelli per cui siamo qui insieme (quelli che insieme non potrebbero stare mai), tutti quei temi sarebbero trascurati, anzi probabilmente non potrebbero essere più trattati. Colleghi, stiamo litigando da mezz'ora, quando tutti sappiamo bene qual è la nostra missione. facciamo riunioni di maggioranza di un Governo di salute pubblica, che non è un governo politico. Lo ripeto ancora una volta, per i malinconici che ancora non l'hanno capito: non è il Governo Conte. Facciamo una riunione di maggioranza e decidiamo insieme quali sono le priorità, ma non possiamo continuare... È il Parlamento, colleghi, mi ricordano che questo è il Parlamento. È il Parlamento che in questo momento sta rappresentando una maggioranza - lo ripeto ancora una volta, a tema di noia - che non potrebbe mai stare insieme su dei temi di carattere generale, ma che ha assunto una missione nei confronti del Paese. Possiamo discutere di tutto, ma lo dobbiamo fare insieme, non a suon di colpi di mano, di botte e di insidie all'interno delle Commissioni, che non rappresentano la natura di questo Governo. Lo ripeto: il tema è molto scivoloso e abbiamo temi molto divisivi sul tavolo. Come voi sapete, io sul punto ho una posizione molto definita, che corrisponde solo a una parte della sensibilità che rappresenta il mio movimento politico. Questo non significa censure, significa condivisione democratica di argomenti all'interno di una maggioranza che ha il primo obbligo di rispettare se stessa e le sue

non qui a fare polemica e a darci mutuamente lezioni di diritti fondamentali, cosa abbastanza mortificante. È vero che questo è il Parlamento, ma ce lo siamo dimenticati tante volte, cari colleghi, proprio voi che adesso lo state dicendo. Quante volte abbiamo fatto passare fiducie, abbiamo fatto "volare" decreti-legge che contenevano ben altri diritti e che gestivano ben altri temi. *(Applausi)*. Abbiamo visto passare come treni in corsa provvedimenti su cui non abbiamo messo mano, non abbiamo messo voce, non abbiamo messo occhi, non abbiamo messo cuore.

Cerchiamo di essere all'altezza di noi stessi e della missione che ci siamo assunti. Siamo un Governo di salute pubblica; comportiamoci come tali. Vediamoci al di fuori di questi consessi e non facciamo polemica. Il Paese non se lo merita e non se lo aspetta da noi.

una Conferenza dei Capigruppo per decidere come andare avanti. *(Applausi)*. Presidente, sono convinto del fatto che il provvedimento possa essere trattato senza che si creino divisioni in Parlamento.

per creare divisioni politiche che giustifichino la collaborazione a sostegno di un Governo che ci vede insieme per gestire la fase emergenziale del Paese.

elementi di drammatizzazione su un tema che credo debba essere affrontato e risolto da questo Parlamento. Credo che il provvedimento possa arrivare in Aula

È un atteggiamento ipocrita perché, se fosse stato approvato quel disegno di legge, Grillo sarebbe stato cacciato a pedate da questo Paese.

*(IV-PSI)*. Io dico che questo disegno di legge può essere benissimo trattato e può essere trovata condivisione tra le forze politiche. Ho letto le proposte di modifica avanzate dalla presidente Valente, che condivido. Ho letto le proposte di modifica presentate dall'onorevole Concia, che condivido. Quindi, se anziché dividersi ideologicamente, ci si siede, ognuno presenta i suoi emendamenti, propone le modifiche e si affronta l'argomento, credo che le forze politiche di questo Paese possano dimostrare maturità

nasce spontanea è chiedersi se questa sia la maggioranza. È questa la maggioranza chiamata a governare il Paese alle prese con la peggiore pandemia della sua storia?

Avete fatto una verifica di maggioranza estemporanea, qui, di fronte a tutti, e avete esibito le vostre divisioni e le vostre contraddizioni. Se questa è la maggioranza che governa il Paese, gli italiani hanno molto, molto di cui preoccuparsi, presidente Alberti

avevamo ragione noi quando dicevamo che non si può stare al Governo con chi la pensa in maniera diversa, se non opposta. Governare con gli opposti non soltanto è inutile, ma è anche dannoso per questo Paese.

Non serve neanche nascondere la polvere sotto il tappeto, invocando riunioni di maggioranza, perché il problema è enorme e non si può nascondere. Noi ritenevamo meglio tornare al voto, avere una maggioranza coesa, una maggioranza con le idee chiare su temi fondamentali come quelli che avete ricordato. E non veniteci a raccontare, come ha tentato di fare anche la senatrice De Petris, che questo è un Governo di scopo, un Governo tecnico. Non esistono Governi tecnici: esistono i Governi. *(Applausi)*. E i Governi sono tutti politici e le contraddizioni che voi oggi avete sottolineato lo dimostrano, se ci fosse bisogno di ulteriori dimostrazioni. Se non siete in grado di governare, se non siete d'accordo, nemmeno minimamente, su temi centrali e di civiltà

però il clima che una parte della maggioranza (mi riferisco, in particolare, al PD e alla sinistra radicale) ha creato è di criminalizzazione per chi osa pensare con la propria testa.

E se domani, una volta approvato il disegno di legge Zan - come spero non accada -qualcuno di noi dicesse che è un diritto fondamentale per un bambino poter pronunciare la parola più bella del mondo, cioè mamma, dovremmo incorrere nelle ire della polizia del pensiero orwelliano della senatrice Cirinnà, che ci ha accusato di squadrismo solo perché esercitavamo il nostro diritto di opposizione in Commissione e in Aula? È questo il sistema che volete creare: una polizia del pensiero che interviene contro chi si ostina a difendere alcuni princìpi fondamentali della nostra Costituzione, della nostra realtà e della nostra civiltà. Questo è il tema fondamentale

Il problema, quindi - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - non è domandarsi quante sono le cose che vi dividono, ma se c'è ancora o se è mai esistito qualcosa che vi tiene insieme,

e che, secondo me, tracollerà sotto il peso di tutto il resto. Questo è uno spettacolo che, purtroppo, il Paese non si merita.

Signor Presidente, vorrei semplicemente riportare il discorso nei giusti termini. Qui non è in discussione il fatto che il Parlamento sia sovrano; il Parlamento può discutere di tutto ciò che vuole. Il problema è un altro ed è stato posto, secondo me correttamente, dal presidente Romeo nella prima parte del suo intervento. Ci troviamo in un momento nel quale non siamo ancora usciti dall'emergenza, abbiamo 400 morti al giorno, i giornali oggi ci dicono che il coprifuoco continuerà fino a luglio.

un problema metodologico e nello stesso tempo politico, ed è il problema che ci ha posto il presidente Draghi. Non entro nel merito della questione; voglio solamente far notare che questo è un tema divisivo e la divisione non è tra oscurantisti, da una parte e illuminati dall'altra. Dubbi su questo disegno di legge sono stati espressi da una femminista storica come Marina Terragni, da una giornalista come Comencini, dall'onorevole Concia e oggi dalla collega Valeria Valente in un'intervista su «Avvenire»,

Questo è il discorso. Nessuno mette in dubbio la sovranità del Parlamento. Quello che si mette in dubbio in questo momento è la responsabilità di una maggioranza. *(Applausi).* PRESIDENTE.

è letteralmente inaccettabile. Il Parlamento è sovrano e può discutere di tutto, anche delle norme e dei disegni di legge divisivi. Detto questo, trovo surreale il teatro che state facendo, che la maggioranza di sinistra e di centrodestra sta facendo sulla legge. Mi pare infatti evidente che voi, mettendo sotto la lente dell'ideologia un argomento così complicato, che state trattando in maniera invece molto superficiale, non facciate altro che tentare di coprire quello su cui invece siete tutti d'accordo. Mi riferisco al fatto di aver delegato tutte le

il Governo vuole spendere i 200 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma ad oggi, ad una settimana da questa data, non sappiamo letteralmente nulla

innalzando i vostri opposti vessilli, che sono del tutto fasulli, per nascondere la verità: siete d'accordo sulla delega dei temi economici che porteranno sciagura al Paese.

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Già approvato in prima lettura alla Camera, il provvedimento si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 capi. L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per trasferirle a un Dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei Ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali in Ministero della cultura. Viene istituito il Ministero della transizione ecologica, che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è denominato Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica, denominato MITE, prevedendo, con una serie di modifiche al decreto suddetto, il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al MITE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema. Le modifiche al citato decreto legislativo riguardano anche l'elenco delle materie attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del nuovo Ministero anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agroenergie. Si specifica che nell'ambito delle materie di competenza del MITE rientrano le autorizzazioni di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili anche se ubicati in mare, oltre che la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare; il ripristino in sicurezza dei siti, la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal Ministero dello sviluppo economico al MITE, rientrano quelle inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del Gestore servizi energetici (GSE l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori in coordinamento con il MISE. Inoltre, sono novellati gli articoli 174-*bis* e 828 del codice dell'ordinamento militare al fine di modificare l'attuale denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale in Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministero della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando altresì la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal Ministero dello sviluppo economico al nuovo Ministero della transizione ecologica. L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. È presieduto dal Presidente del Consiglio, e in sua vece dal Ministro, e approva il piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare.

sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo a tal fine novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone inoltre l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel citato decreto legislativo 300 del 1999 gli articoli 54-*bis* e 54-*quater.* A tal fine l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stato riconosciute. L'articolo 8 reca una serie di disposizioni concernenti

anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo istituito Comitato interministeriale. Il gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza Covid, viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Conseguentemente, le risorse del fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. i regolamenti del 2021 di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, nonché del lavoro e delle politiche sociali, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dalla legge n. 400 del 1988, all'articolo 17, che prevede che i regolamenti governativi siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano gli aspetti riguardanti la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

dopo lo spettacolo offerto questa mattina dalla maggioranza, come esponente di Fratelli d'Italia sono ancora più fermo nelle convinzioni che il partito ha espresso in lungo e in largo. di questo Governo ci siamo soffermati più volte, evidenziandone le contraddizioni, l'inadeguatezza e le storture. Questo provvedimento sul riordino

delle carenze che ho esposto in premessa. È un provvedimento che, lungi dall'essere propedeutico al raggiungimento di una maggiore efficienza amministrativa, rappresenta lo strumento, realizzato con grande capacità di equilibrismo politico, per raggiungere i *desiderata* e le esigenze dei partiti che fanno parte di questa maggioranza. Ne sono la testimonianza concreta le sorprendenti e fantasiose formule lessicali utilizzate

innovative quanto vuote di concretezza, ma altrettanto strumentali - come dicevo - per accontentare le esigenze di retorica e di posizionamento dei partiti che compongono questa eterogenea maggioranza. In tutto questo contesto spicca un'assenza clamorosa: mi riferisco alla mancanza del Ministero dello sport. Come Fratelli d'Italia si siamo soffermati più volte su questa assenza, resa ancora più grave

quanto e come potranno essere considerate le riaperture in ordine al possibile raggiungimento di una situazione a regime delle economie delle delle singole attività sportive e dei singoli impianti sportivi. Ci troviamo di fronte ad aperture a singhiozzo, limitate a un massimo del 30 per cento, di fronte a un'unica certezza: il 100 per cento dei costi e l'impossibilità di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario. Pertanto, parlare di aspetti burocratici, parlare di un Ministero potrebbe sembrare fuori luogo in questa circostanza e offensivo nei confronti degli organismi sportivi, delle società e delle associazioni che sono in sofferenza. Non lo è, perché purtroppo questo risultato è figlio di una cultura inesistente nel nostro Paese, della mancanza di considerazione per il comparto dell'impossibilità di capire quanto questa materia sia importante per le dinamiche di crescita del Paese. Sono processi che hanno portato non solo all'abolizione del Ministero dello sport, ma anche all'insussistenza dei provvedimenti adottati in questo periodo dal Governo, che purtroppo hanno lasciato inalterate le risposte: mi riferisco sia al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia al decreto sostegni.

dal consolidamento delle medaglie olimpiche alla costruzione di un'Italia sportiva. Questo è l'obiettivo per il quale dobbiamo arrivare a invertire la tendenza, che poi si riflette drammaticamente anche nelle parole dei nostri governanti. Siamo passati dalla considerazione delle attività sportive,

alla situazione italiana, anche all'interno del contesto europeo, cercando di capire come negli altri Paesi viene vissuto il rapporto con il mondo dello sport. In tutti i Paesi europei - lo sottolineo: tutti - esistono autorità governative, a volte espressione di un Ministero, a volte comunque espressione di altre autorità pubbliche, che si occupano di sport. Solo in Italia questo non è mai accaduto. È vero che nel passato ci sono stati dei Ministeri che si sono occupati di questa materia, tutti rigorosamente senza portafoglio e con competenze limitate. Cos'è accaduto in Italia, nel corso di questi anni? Nel Dopoguerra, purtroppo, il nostro Paese, nell'intento di tutelare e legittimare l'operato del CONI, gli ha però delegato tutte le incombenze di carattere sportivo. Ciò ha prodotto un disinteresse da parte dello Stato, il CONI se l'è comunque cavata egregiamente, ma non ha potuto fare nulla per individuare il modo attraverso cui cui far crescere, all'interno del Paese, una consapevolezza, rispetto al mondo dello sport, che passasse attraverso l'affermazione di due dei pilastri che consentono la crescita di una cultura sportiva, ovvero il rapporto con la scuola e quello con la salute. In mancanza di questi due pilastri, non è mai stato possibile sviluppare, per mancanza di interlocutori, un ragionamento di carattere strategico. ha comunque supplito alle carenze statali, perché fino a quando è stato autonomo finanziariamente, ha potuto dare delle risposte, anzi era lo sport che dava soldi allo Stato italiano e non viceversa, e c'era comunque la possibilità,

ha iniziato però a smantellare progressivamente questo sistema, che - lo ripeto - comunque funzionava. Come lo ha smantellato? Da questo punto di vista, le responsabilità della sinistra sono enormi. Mi riferisco al primo Governo Prodi, all'allora ministro Veltroni che, nell'andare a regolamentare alcune norme riguardanti la vita dell'ordinamento sportivo italiano, introdusse un principio che, arrivando ai giorni nostri, ha prodotto poi degenerazioni: la lucro all'interno del mondo dello sport. Fino ad allora la mancanza del fine di lucro era stato un fondamento, un pilastro, che aveva permesso in termini di mutualità di dare risposta a tutto un sistema. Per colpa della sinistra, per colpa di Veltroni, l'introduzione del lucro

una corsa al lucro, un forte indebitamento e una situazione per la quale i club professionistici si apprestano ora a trovare nuove soluzioni. Ci sono ovviamente le responsabilità anche delle istituzioni sportive, ma non è questa la sede per parlarne. È curioso e singolare, forse anche imbarazzante, il silenzio del CONI, ma ad oggi quello che dobbiamo fare - ed è il male minore, ne parlavo poco fa con il presidente La Russa - è difendere le istituzioni sportive nonostante le grandi responsabilità. responsabilità. Avviandomi a concludere, c'è necessità quindi di invertire la rotta, ma per farlo dobbiamo assolutamente partire dalla madre di tutte le leggi italiane, dalla Costituzione. Sino a quando non troveremo il modo per introdurre lo sport come diritto all'interno della Costituzione italiana, non riusciremo mai a creare le basi per andare a

il decreto-legge di cui stiamo discutendo inerisce al riordino delle competenze, delle funzioni e dell'organizzazione di più Ministeri.

L'illustrazione generale del provvedimento è stata fatta molto bene dal collega relatore che mi ha preceduto. Come componente della 13a Commissione del Senato intendo fare però alcune riflessioni sull'articolo 2

c'è il trasferimento delle competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico al nuovo Ministero, oltre ad una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. In questo contesto si inseriscono impostazioni diverse su competenze che già erano in capo al vecchio Ministero. Non c'è soltanto un trasferimento di funzioni, quindi, ma anche le competenze che erano già in capo al vecchio Ministero vengono declinate declinate in modo diverso e mi riferisco in particolare al riconoscimento, finalmente - era ora che vi fosse, a mio parere, anche se troppo leggero - di un ruolo per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che precedentemente non era presente. Sulle importanti tematiche ambientali, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'agricoltura non hanno mai avuto modo, negli ultimi anni, di trovare soluzioni congiunte o comunque su tematiche importanti come quella delle gestioni, ad esempio quella faunistica, ha sempre prevalso una linea protezionistica del Ministero dell'ambiente. Oggi credo che non sia più così, anche perché l'estremismo protezionista di chi ha gestito il Ministero dell'ambiente nello scorso Governo non c'è più e quindi credo che ce lo possiamo dimenticare Appare quindi in un decreto-legge, per la prima volta, un segnale di raccordo tra i ruoli dei due Ministeri e questo è importante perché, com'è noto, la più la più grande parte del territorio del nostro Paese non è città, né zona urbanizzata, bensì costituisce un importante polmone che tutti vogliamo preservare e che magari troppo spesso ci dimentichiamo che esiste.

quando questo è avvenuto per colpa della parcomania estremista cui abbiamo assistito in Italia, i risultati hanno portato al degrado ambientale: il principio dell'abbandono dell'ambiente a se stesso, perché l'uomo non avrebbe diritto o titolo di metterci piede alla fine, se questo ambiente non è gestito, porta cioè al degrado ambientale. Diventano quindi ancora più fondamentali; soprattutto oggi, la presenza e l'intervento ragionevole dell'uomo. La visione di questo fattore in un'ottica agro-forestale è diversa rispetto a quella di chi la vuole vivere in una ambientale, orientata unicamente ai sentimenti e dimenticando la razionalità.

in una sentimentale, alla quale abbiamo assistito - non c'è ombra di dubbio che spesso nella gestione di queste tematiche piuttosto che la razionalità abbia prevalso la sensibilità *tout

per riconoscere l'importante ruolo di chi mantiene sano l'ambiente naturale e che oggi è osteggiato dall'ambientalismo di salotto, che ogni tanto emerge anche all'interno di quest'Aula. Totale rispetto va a quei pochi che gestiscono e mantengono vivo e sano l'esteso territorio del nostro Paese.

Un ambiente sano, naturale e ben gestito consente all'uomo di prelevare aria, acqua, vegetali e animali. Lo diremo all'infinito: per noi anche l'uomo fa parte della biodiversità.

la grande novità lanciata dal MoVimento 5 Stelle per la rivoluzione verde del nostro Paese e raccolta dal neonato Governo. Il lessico della transizione ecologica non deve implicare una conoscenza compiuta di una meta già stabilita; piuttosto, deve indicare un continuo cammino verso una piena ecosostenibilità dei processi antropici, sulla base di un cambiamento profondo del pensiero umano. Finora abbiamo inseguito gli accecanti bagliori del PIL, che hanno condannato il pianeta al soffocamento. Non vi sembra sia oramai giunta l'ora del progetto Bes, il benessere equo e sostenibile come marcatore di quello umano? Per tale cambio di paradigma socio-economico occorre una transizione verso il vero progresso. La scienza ci verrà in soccorso, ma bisognerà sempre lanciare il cuore oltre ogni ostacolo che troveremo sulla nostra strada, per poi saltare tutti insieme. quindi auspicabile aggiungere nella sostanza un aggettivo: transizione ecologica e solidale. Forse sarebbe ancora più appropriato parlare di conversione ecologica, così come, con geniale intuizione, fece un trentennio fa l'indimenticabile Alex Langer, ecologista e sostenitore del *lentius, profundius, suavius*, più lento, più profondo e più dolce, le tre parole chiave dell'ecologia. Poi il concetto è stato ripreso, in prospettiva religiosa, dagli ultimi tre pontefici e superbamente da Francesco nella sua enciclica «Laudato si'». Conversione ecologica è un'espressione che ha un risvolto soggettivo, etico, e uno oggettivo, sociale. È il cambiamento del nostro stile di vita, del nostro lavoro, dei nostri consumi e del nostro rapporto con gli altri e con l'ambiente. La conversione è ecologica perché tiene conto dei limiti dell'ambiente in cui viviamo, principalmente temporali: sia perché siamo mortali in un mondo che ci sopravvive, toccando quindi la nostra più intima sfera esistenziale, sia perché ci ricordano che non possiamo consumare più di quello che la natura è in grado di produrre, né inquinare più di quanto l'ambiente riesce a rigenerare.

per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica, per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari. Al Mite sono attribuiti i vecchi compiti del Mattm, alcuni compiti del Mise e nuovi compiti in tema di economia circolare, pianificazione strategica per la riduzione delle emissioni inquinanti, trasporti sostenibili, produzione e mercato energetico, nonché bonifica dei siti inquinati. Va bene dunque il ripensamento del Ministero in termini di organicità, semplificazione ed efficientamento delle politiche nazionali in campo energetico. bene anche l'attribuzione delle funzioni per il contrasto ai cambiamenti climatici, nonché per risparmio ambientale, migliore qualità dell'aria e finanza sostenibile. Questi sono i tre pilastri da cui partire per ripensare i modelli economici a cui siamo stati abituati sin dalla prima rivoluzione industriale. Perché qualcosa davvero cambi, è necessario che economia e ambiente diventino due facce della stessa medaglia.

tutti sappiamo che non può esserci sviluppo economico senza tutela dell'ambiente, perché esso deve diventare ecosostenibile e durevole. Perché ciò sia, occorre accrescere anche la tutela del territorio e del mare. Come si potrebbe parlare di transizione ecologica con un territorio inquinato, abusato, insicuro, non sufficientemente monitorato e conosciuto? Il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo, i corpi idrici interni, il mare, le coste, le terre dei fuochi, i parchi naturali e la biodiversità dovranno essere il punto di partenza di ogni attività. In un Paese geologicamente fragile, il Mite deve attuare con organicità i necessari interventi strategici per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi naturali.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 si può realizzare una segreteria tecnico-amministrativa per la programmazione, il monitoraggio e l'implementazione del Piano per la transizione ecologica, che diventi un punto di riferimento per istituzioni, agenzie governative, enti di ricerca e privati. Per la programmazione degli interventi - e non solo in emergenza - si può creare un modello di *governance* che impieghi le migliori competenze del nostro Paese a livello nazionale e locale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Per gestire al meglio le risorse a nostra disposizione (penso al Piano nazionale di ripresa e resilienza) si possono attuare nuovi modelli operativi che garantiscano efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza nell'impiego delle risorse finanziarie statali ed europee per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Basta con inutili e dannosi ritardi per la realizzazione delle opere, non abbiamo più tempo per le scuse. Sia il Mite la soluzione al nodo gordiano di tutte le onerose politiche programmate per la transizione ecologica. Siccome Siccome la meta della transizione ecologica è dinamica, non la si può racchiudere in un improbabile algoritmo, date le molteplici variabili del sistema (alcune delle quali etiche), altrimenti il rischio è che per correggere gli errori ne commettiamo altri, magari anche peggiori. Le centrali nucleari, sono un esempio, come i magici inceneritori che fanno sparire le ecoballe. È il motivo per cui preferisco la conversione ecologica: stabilire la luce che deve illuminare l'azione politica, la ricerca scientifica, l'ecosostenibilità, la giustizia, la libertà, la condivisione e la solidarietà. Sulla base di questi capisaldi si dovrà sviluppare tutto il potenziale politico e innovativo di questo Ministero. Buon lavoro, ministro Cingolani. Infine, vorrei ricordarvi che domani, 22 aprile,

credo che la decisione di riordinare i Ministeri sia stata saggia e rispondente alle necessità del Paese. In particolare, è emblematica la creazione del Ministero del turismo, che risponde a una doppia esigenza di buon senso e necessità. buon senso perché non era pensabile che l'Italia, che vanta senza dubbio il più grande patrimonio artistico, architettonico e naturale al mondo, con le sue migliaia di chilometri di spiaggia, le sue celebri montagne e le città d'arte che tutto il mondo ci invidia, non avesse un Ministero dedicato al turismo, settore che da solo rappresenta una fetta importante del nostro PIL. Parlo anche di necessità perché ora più che mai, dopo la terribile scure agli introiti turistici causata dalla pandemia, il settore ha bisogno della massima concentrazione di sforzi da parte del Governo, per trovare soluzioni alla crisi e strategie giuste per il rilancio. Pensiamo solo a cosa ha rappresentato il 2020 per le migliaia di aziende italiane che operano nel settore turistico, dagli alberghi ai ristoranti, ai *tour operator*, ai *bed and breakfast*, alle guide turistiche: molti miliardi di euro di ricavi sono stati persi in un solo anno e c'è un numero di aziende fallite e di persone che hanno perso il posto di lavoro che forse ancora non abbiamo nemmeno calcolato. Il primo trimestre del 2021 non ha certo rappresentato un'inversione di tendenza; anzi, se possibile, ha ulteriormente peggiorato il quadro, visto che tutto il comparto che lavora sulla stagione sciistica invernale ha visto il fatturato ridursi praticamente a zero. Solo nei prossimi mesi verranno tristemente a galla gli effetti drammatici a livello economico e occupazionale di questo lungo e buio anno di pandemia. Il coronavirus ha lasciato dietro di sé una profonda scia di distruzione dal punto di vista delle attività imprenditoriali e dei posti di lavoro che garantivano; per rinascere in fretta dalle ceneri servono programmazione e una strategia complessiva. Trovo quindi sensato e logico che un settore vitale per la nostra economia come quello del turismo abbia un Ministero dedicato. Le competenze erano troppe e gli ambiti di intervento troppo vasti perché fosse unito ai beni culturali. Per quanto riguarda invece la variazione di denominazione dei Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, credo che sia giusto dare una maggiore attenzione al rispetto e alla tutela dell'ambiente che ci circonda. Lo dico da senatore Lo dico da senatore proveniente da un piccolissimo Comune montano della Provincia di Torino, di nemmeno 1.000 abitanti, dove l'attenzione alla salvaguardia del territorio non è una politica, ma un modo di vivere da secoli. La cura per l'ambiente che ci circonda e il miglioramento dell'aria che respiriamo non possono che rivestire un ruolo fondamentale nelle politiche di... ...evitando gli eccessi, al contempo, anche di certe iniziative di facciata, che hanno un'eco sui *media* inversamente proporzionale agli impatti pratici sull'ambiente.

È facile fare l'ambientalista per chi ha il SUV elettrico da 50.000 euro e l'attico in centro storico; lo è molto meno per l'operaio o l'artigiano con un'utilitaria diesel e un appartamentino in periferia, che si deve barcamenare tra le esigenze di lavoro, il traffico sempre più congestionato e i divieti di circolazione. Mi auguro che il Ministero per la transizione ecologica operi nel solco di quella concretezza, praticità e buon senso che finora hanno contraddistinto l'opera del Governo Draghi, che in questo senso ha rappresentato, sin da subito, un netto punto di svolta rispetto all'esperienza precedente, improntata alle dirette Facebook, ai monopattini e ai banchi a rotelle. Dividere il tempo in pochi minuti rende difficile l'intervento, per cui la ringrazio per averlo sintetizzato,

che consenta di strutturare una nuova economia basata sull'ambiente, con nuove imprese e nuovi posti di lavoro, ma soprattutto meno lavoro e affrontato in maniera migliore. la pandemia ci ha insegnato qualcosa, colleghi, è proprio che, se sta bene l'ambiente, stiamo bene anche noi. Troppo in questi anni è successo senza che ci fosse un approccio serio ed ecologico al percorso del nostro Paese.

che ha portato alla produzione di 2 milioni di biciclette in più (quasi il 20 per cento in più) rispetto al 2019. Sono cifre molto importanti nel periodo di crisi che abbiamo affrontato nel 2020.

Altri argomenti che abbiamo portato avanti in questo momento, sempre nel solco della transizione energetica, sono le comunità energetiche, che sono un punto basilare su cui abbiamo investito

Tutti questi provvedimenti vanno nel percorso dell'efficienza energetica, ma il paradigma è completamente differente. Bisogna diminuire il consumo e dare un ciclo vitale a quanto si produce.

Stiamo vivendo un momento veramente drammatico per questo settore, che oggi soffre in maniera veramente importante. Rappresenta il 13,2 per cento del PIL del nostro Paese e in alcune Regioni - tengo a dirlo - addirittura il 25. È davanti a una difficoltà drammatica e nel 2020 ha perso oltre 60 miliardi. Il 2021, purtroppo, non è iniziato molto bene per il primo *lockdown* che abbiamo dovuto affrontare. quindi tanto terreno da recuperare per questo Ministero, che - lo ricordo a tutti - è stato abrogato nel 1993 in seguito a un *referendum* abrogativo, purtroppo sotto l'alone del cancellato finanziamento pubblico ai partiti, cui noi abbiamo rinunciato, mentre molti altri hanno trovato il modo di reintercettare quei soldi.

e il comparto enogastronomico che hanno possibilità di ricevere attenzione in maniera molto più particolare. Il Ministero avrà una cabina di regia importantissima in questo momento. Purtroppo, per anni abbiamo venduto il turismo in maniera capillare, senza far capire la grandezza del nostro Paese e l'unicità della meta turistica.

Signor Presidente, faccio un appello soprattutto al nuovo Ministro e, in particolare, al nuovo Governo. L'anno scorso il presidente Conte in questo periodo spinse tantissimo e a gran voce

andate in vacanza ha scelto l'Italia. Potevano scegliere anche altri Paesi, ma sono rimaste per aiutare gli imprenditori e il nostro territorio e per un'economia più sostenibile. Faccio a

Signor Presidente, colleghe e colleghi del Senato, conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, mette al centro l'importanza del neonato Ministero della transizione ecologica, ecologica, che riunisce il vecchio Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, accorpando di fatto le funzioni che lo caratterizzavano con quelle relative alla politica energetica e mineraria proprie del Personalmente guardo con fiducia a questo Ministero, perché, rispetto al precedente, oltre alle funzioni di tutela dell'ambiente, ha anche quelle relative alla sua valorizzazione senza trascurare l'aspetto dell'ecosostenibilità. quindi una nuova visione integrata e trasversale, che prevede il concetto di ambiente nella sua più ampia accezione, che è centrale e cruciale, in quanto dovrà consolidarsi un approccio non limitato solo alla protezione e alla custodia, ma volto totalmente allo sviluppo sostenibile dei territori. La visione integrata di cui ho appena parlato può comprendere l'agricoltura e, con essa, il turismo, due realtà complementari e inscindibili, capaci di creare opportunità per chi vive i territori tutto l'anno e per chi li sceglie come luogo di riposo e vacanza. La Provincia in cui vivo, Belluno, è un esempio concreto per capire come vi sia la possibilità di tutelare l'ambiente, di valorizzarlo e di renderlo una opportunità. Tutti voi conoscete senza dubbio la bellezza delle Dolomiti, dei paesaggi costellati da malghe e pascoli, nonché dei preziosi e curati boschi e dei laghi. Tutto questo patrimonio è ancora lì, integro e visibile: si è tramandato nei secoli grazie alla capacità dell'uomo di vivere in sintonia con la natura. Da sempre l'essere umano ha potuto godere dei prodotti montani, dedicandosi all'agricoltura, all'allevamento, alla silvicoltura e alla conseguente lavorazione del legno. Questo splendido meccanismo si è purtroppo inceppato una quarantina d'anni fa, quando la forte industrializzazione a valle ha mutato l'equilibrio tra uomo e montagna. Si è verificato un graduale abbandono della cura dei territori alti, con una conseguente espansione non controllata dei boschi, causa prima del dissesto idrogeologico. Negli ultimi anni la Regione Veneto, in sintonia con le direttive europee, ha finanziato, attraverso progetti importanti, la ripresa dell'agricoltura montana. Quest'opportunità, legata poi alla crisi del 2007, ha fatto sì che molti giovani siano ritornati alla cura della terra, valorizzandone i prodotti e creando un circolo virtuoso, sia per la distribuzione sia per la consumazione. L'impegno, infatti, è quello di proporre i prodotti anche nella ristorazione, che molto spesso da noi è stellata, a riprova della loro qualità. Un altro aspetto Un altro aspetto importante, da non sottovalutare e da prendere seriamente in considerazione, è quello della cura dei boschi e della conseguente filiera del legno. In questi mesi di crisi sono emersi aspetti negativi: da gennaio, per esempio, i prezzi dei cosiddetti prodotti segati del legno, che importiamo dall'Austria, hanno subito rincari che sfiorano il cento Ancor più penalizzante, però, è la difficoltà a trovare fornitori che garantiscano le consegne in tempi adeguati. Ciò mette in difficoltà le nostre industrie dell'arredo e degli imballaggi, il settore edile e altro.

Vorrei però ricordare che la gestione sostenibile dei boschi è stata ideata dal Repubblica marinara di Venezia, che necessitava di tanto legno: tutta la città è costruita su tronchi di legno per la solidificazione della laguna, e pensiamo a tutte le navi necessarie per l'attività sia mercantile sia bellica. Ebbene, Venezia, che aveva grandi foreste nel Nord-Est e in territorio sloveno e croato, si preoccupava che, per ogni albero tagliato per le proprie esigenze, ne fosse piantato un altro. Questo le ha permesso di andare per i mari e contemporaneamente di far arrivare fino a noi le foreste ancora integre. Il mio auspicio, quindi, è che si ritrovi una particolare attenzione verso tutti gli argomenti che ho appena elencato, ritornando, oltre che all'agricoltura di montagna, che già è una bella realtà, alla silvicoltura, l'agricoltura del bosco, con un rilancio della filiera del legno con la lavorazione *in loco* dei tronchi e dismettendo l'attuale pratica che prevede la lavorazione in Austria e la rivendita nei mercati degli Stati Uniti. Solo così potremo salvare ambiente e industrie ed evitare uno spopolamento della montagna che ormai sembra inesorabile.

le problematiche legate alle espressioni "questione ambientale" e "cambiamento climatico" stanno velocemente diventando centrali di fronte alle emergenze sempre più frequenti provocate dai danni apportati agli ecosistemi terrestri e marini per effetto delle attività umane, dovute a modelli industriali ormai non più sostenibili per preservare gli attuali equilibri che regolano l'ambiente e il clima del nostro pianeta. Il cosiddetto Earth overshoot day (EOD), letteralmente il giorno del superamento terrestre, nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal nostro pianeta nell'intero anno, viene anticipato periodicamente. Si stima che, procedendo con questo ritmo, nel 2050 l'umanità consumerà ben il doppio di quanto la Terra riesca a produrre. questa una situazione che diventerà insostenibile in un futuro non lontano per le condizioni di vita e di salute delle persone. A livello internazionale, gli Stati hanno iniziato a prendere coscienza che il tempo a disposizione per intervenire e invertire questa tendenza è sempre meno

A questi accordi dobbiamo aggiungere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per uno sviluppo sostenibile e il *green deal* europeo, avente l'obiettivo di conseguire la cosiddetta neutralità climatica, ossia l'azzeramento delle emissioni nette di gas effetto serra entro il 2050 nell'area dell'Unione europea come primo continente al mondo a raggiungere tale importante risultato. *(Applausi)*. di questa mattina che l'Unione europea ha raggiunto un accordo con l'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030. I dati dell'Ispra dicono che il calo di CO2 dell'Italia rispetto al 1990 è ad oggi circa il 17 per cento. Ciò significa che l'Italia deve ridurre del 38 per cento le sue emissioni in meno di nove anni. Da questo contesto internazionale si capisce che le sfide ambientali che il nostro Paese deve affrontare sono molto complesse e riguardano ogni settore dell'economia. I cambiamenti che definirei epocali, la produzione di energia, la mobilità pubblica e privata, la produzione di alimenti e la costruzione di infrastrutture, di immobili civili e industriali devono

implementando processi industriali per creare prodotti o servizi che abbiano un impatto positivo sia sull'uomo sia sull'ambiente. Tutto ciò va nella direzione della transizione ecologica verso il punto d'arrivo della cosiddetta economia circolare, in quanto il prodotto viene validato con cinque aspetti: la salubrità dei materiali e il loro riutilizzo, la gestione delle risorse idriche, l'utilizzo di energia rinnovabile e l'equità sociale. Per tutti questi motivi, il Ministero della transizione ecologica diventa centrale e indispensabile per l'attuazione degli obiettivi imposti dai suddetti accordi internazionali, soprattutto il *green deal* europeo, nonché per la realizzazione del Next generation EU, che porterà al nostro Paese 209 miliardi

tema della transizione ecologica è centrale per noi del MoVimento 5 Stelle e non a parole, ma con i fatti. Basta guardare al superbonus del 110 per cento e alle comunità energetiche, che vanno nella direzione dell'efficientamento energetico, della mitigazione ambientale e, contemporaneamente, del benessere sociale, verso la democratizzazione dell'energia, compresa la riduzione del costo finale per gli utenti. Tornando al riordino dei Ministeri, altro importante passo in avanti è l'introduzione del Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, proprio per le sfide

stimolare il passaggio a nuove tecnologie ecosostenibili e rendere quanto più accessibile e burocraticamente semplice la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali In tale contesto, sarà fondamentale avere una migliore digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, che sia realmente efficiente e fruibile dai privati e dalle imprese, affinché sia possibile rilanciare molte attività economiche e stimolare l'ingresso di nuovi imprenditori, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro. Con un efficiente e veloce sistema di accesso alla rete Internet in tutto il Paese, non solo nelle grandi città, ma anche nei paesi più remoti d'Italia, cercare di creare opportunità per un tessuto economico e imprenditoriale nel quale fino ad oggi ci sono stati abbandono e desertificazione. Occorre creare strumenti e opportunità per i tantissimi piccoli imprenditori, agricoltori e artigiani che rappresentano uno dei punti di forza dell'intera economia italiana, affinché possano sviluppare le proprie capacità imprenditoriali, aumentando la loro ricchezza personale e quella dell'Italia in generale. Il nostro Paese è chiamato ad affrontare le sfide derivanti dallo sconvolgimento climatico con consapevolezza e conoscenza. Pertanto, l'innovazione tecnologica e digitale e la transizione ecologica dovranno essere considerate primarie nei prossimi anni, anzi, già da oggi, giacché la scadenza del 2050 e, ancor prima, quella sono, in termini di protezione dell'ambiente e del benessere collettivo, iniziando dalla salute pubblica, da considerare praticamente dietro l'angolo. *(Applausi)*.

al nostro esame, non è semplicemente un decreto Ministeri, ma in realtà è il modo in cui il Governo ha dato le prime risposte ai cittadini. Mi riferisco in primo luogo alla creazione di un Ministero del turismo. In questi mesi ho avuto modo di ascoltare molti operatori del settore turistico: sono disperati. La crisi pandemica, che ha causato perdite drammatiche a tutta la nostra economia, ha completamente devastato il settore turistico. I dati sono allarmanti e gli interventi messi in campo nella prima fase dell'emergenza sanitaria sono risultati inadeguati e insufficienti. Il 2020 si è chiuso con una perdita 236 milioni di presenze, con un calo medio di oltre il 54 per cento rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80 Il 2021, come purtroppo era immaginabile, è iniziato mostrando un ulteriore peggioramento, anche a causa del perdurare del blocco dei flussi internazionali, del divieto di spostarsi da una Regione all'altra e delle limitazioni alle attività e ai servizi che caratterizzano i viaggi per vacanza e per lavoro. Ci sono attività devastate da questa crisi. Oltre alle agenzie di viaggio e alle imprese del settore degli autoservizi, che hanno avuto un periodo difficilmente superabile,

La nascita del Ministero del turismo è un segnale chiaro per sottolineare l'importanza del ruolo che il Governo riconosce al turismo, per offrire un sostegno concreto agli sforzi delle imprese che oggi soffrono che, al termine della pandemia, saranno chiamate a confrontarsi con un'agguerrita concorrenza internazionale. Il nuovo Ministero, che è inserito nella visione complessiva del piano di Governo esplicitata in questo provvedimento, cioè nella volontà di procedere con risolutezza verso la digitalizzazione del Paese, può avere grandi prospettive. Penso a quanto sarebbe importante sostenere lo sviluppo in chiave sempre più digitalizzata delle imprese che operano nel settore turistico, alla semplificazione burocratica degli adempimenti cui le aziende del settore devono sottostare, all'utilizzo di nuove tecnologie in questo campo, all'attivazione di percorsi formativi indirizzati alla conoscenza e all'utilizzo degli strumenti digitali. Le sfide sono molte e il provvedimento in esame ha cercato di spiegare qual è l'organizzazione che il Governo si è voluto dare per affrontarle.

Governo, onorevoli colleghi, oggi discutiamo un provvedimento per il riordino delle attribuzioni dei Ministeri che si inserisce in una logica fondamentale di questo Governo, quella cioè di affrontare un periodo terribile della nostra storia nazionale e globale.

ritengo fondamentale perché, come è già stato detto in quest'Aula, questo settore della nostra economia, ma anche della nostra storia e - oso dire è quello che sta pagando il prezzo maggiore da poco più di un anno a questa parte. Pertanto, sperando di riuscire a venir fuori da questo terribile periodo, è fondamentale che ci sia un Ministero dedicato a questo straordinario comparto della nostra economia. L'altro aspetto che ritengo fondamentale è l'aver accorpato

dell'umanità abbiamo stravolto il nostro pianeta e, come ricordava qualcuno poco fa, domani ricorre la celebrazione della giornata della terra. Lo abbiamo stravolto come non è mai accaduto in milioni di anni e lo abbiamo fatto fondamentalmente

avere spostato il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nelle competenze del Primo Ministro o, in sua vece, del Ministero della famiglia. Abbiamo un dovere fondamentale, che è quello di lasciare questo mondo ai nostri figli in condizioni migliori di come l'abbiamo trovato. Signor Presidente, membri del Governo,

Prova ne sono i tanti emendamenti presentati sia alla Camera che in questa sede, tutti diretti a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei Ministeri. Purtroppo il corso dell'*iter* e la conclusione di questa prima fase che ha portato il testo in seconda lettura al Senato ci ha in gran parte deluso; questo non per la bocciatura quasi totale dei nostri emendamenti, ma per la logica che che abbiamo visto guidare questa riorganizzazione, che ci è parsa più da manuale Cencelli che non ispirata a criteri di efficienza, a causa della spartizione delle competenze e dei riequilibri dei pesi e contrappesi di ogni singolo Ministero a seconda del riferimento politico del Ministro. Penso in particolare alle molte competenze attribuite al Ministero della transizione ecologica, che ha assorbito deleghe importanti, che erano fino ad oggi di competenza del Ministero dello sviluppo economico; deleghe tali che potrebbero generare problemi di efficienza, tenuto conto che dovrà occuparsi non solo dell'importante settore delle energie, ma anche dei consorzi di bonifica, di dissesto idrogeologico e di nucleare, ossia tutta una serie di competenze che hanno infatti già costretto a prevedere comitati e cabine di regia che riteniamo però di difficile gestione. Forse il pensiero era più quello di depotenziare il Ministero dello sviluppo economico che non di ottimizzare quello della transizione ecologica. D'altra parte, il Ministero della transizione ecologica, che ha sostituito - come sappiamo - il Ministero dell'ambiente, con un nome che già identifica un aspetto a mio è l'ultimo baluardo della politica grillina; anzi, più che l'ultimo baluardo direi l'ultima scusa per giustificarne l'ingresso in questo Governo. dal «mai con Salvini» al «mai col partito di Bibbiano»; dal «mai con Berlusconi» al «mai con il banchiere Draghi»; insomma, occorreva una foglia di fico per giustificare l'ennesimo voltafaccia di un movimento che ha tradito tutto pur di rimanere incollato alle sedie del potere. Il Ministero della transizione ecologica era il giusto prezzo, ma questo è un aspetto che gli elettori sapranno valutare. Quello che ci preoccupa, invece, sono le sorti del Paese, pensando alle politiche energetiche, elemento fondamentale per il sistema economico nazionale. Tutto questo è messo in mano al partito del «no»: no al TAP, no alle trivelle, no alla TAV; no a tutto, ma sì alle poltrone. altro aspetto che ci ha profondamente deluso è la cancellazione del Ministero dello sport, ma abbiamo già visto - come il collega senatore Barbaro ha colto meglio di me - l'aspetto negativo di tale scelta. Mi permetto solo di sottolineare come questa scelta sia sbagliata anche alla luce di quanto sia mancata una giusta attenzione ad un settore profondamente in crisi a causa delle scelte fatte da questo Governo per contenere il contagio da Covid, ma è inopportuno anche in vista degli importanti appuntamenti di carattere mondiale che vedrà lo sport italiano impegnato in importanti sfide nel prossimo futuro. Un aspetto invece in parte positivo lo ritroviamo nella costituzione del Ministero del turismo. Dopo gli ultimi rimpalli da un Ministero all'altro, che ha visto il turismo trattato come una semplice delega da attribuire a questo o a quell'altro Ministero, finalmente si è capito che questo settore è fondamentale per l'intera economia nazionale e che doveva avere un riconoscimento e un'attenzione propria. Voglio ricordare, in questa sede, le battaglie di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, che hanno sempre spinto in questa direzione, presentando anche disegni di legge che intervenivano in maniera determinante sulla ripartizione delle varie competenze, anche nei confronti delle Regioni.

La verità è che nella maggioranza esistono due correnti di pensiero, forse anche più di due, contrapposte e difficilmente conciliabili: da una parte c'è chi vorrebbe investire e costruire e dall'altra chi invece si oppone a tutto. infatti parlando di infrastrutture fondamentali per il Paese - ferroviarie, stradali, aeroportuali e marittime - e dei collegamenti vitali per la vita economica e sociale della Nazione. Non possiamo giocare solo con i titoli, senza dare sostanza.

risorse, per garantire il servizio, mantenendo la sicurezza sanitaria a bordo. Da mesi stiamo denunciando che il trasporto pubblico è uno dei potenziali luoghi di trasmissione del virus e non lo dice Fratelli d'Italia, ma i Nuclei (NAS). Se la risposta del Governo è introdurre la mobilità sostenibile nella denominazione del Ministero, ci sembra un po' poco, non ci basta e non è sufficiente. infine, signor Presidente, un tema che ci sta particolarmente a cuore, su cui da tempo abbiamo presentato dei disegni di legge, sia al Senato, sia alla Camera dei deputati, a prima firma del presidente Giorgia Meloni. Da tali disegni di legge abbiamo estrapolato degli emendamenti, che abbiamo presentato al esame e che, sostanzialmente, chiedono la costituzione di un Ministero del mare. Si tratta, purtroppo, di un tema spesso ignorato e a volte relegato ad una semplice delega, che fa torto ad un settore strategico per la Nazione. L'Italia è infatti una piattaforma naturale in mezzo al Mediterraneo. Questa sua posizione strategica ha da sempre condizionato la nostra storia, che è infatti legata al mare e alla navigazione, basti ricordare le Repubbliche marinare e il nostro primato come grandi navigatori ed esploratori.

e circa il 25 per cento nel Mediterraneo e l'Italia si trova ad avere sempre di più una posizione geografica fondamentale e privilegiata. Eppure questo vantaggio non è stato sfruttato, perché non esiste una politica capace di comprendere e sviluppare il ruolo geopolitico dell'Italia, né di comprendere quanto la *blue economy* è e potrebbe essere, se ben supportata, una risorsa straordinaria per la nostra nazione. nazione. Questa miopia, che si riflette in ritardi infrastrutturali e burocratici, non solo ci fa perdere numerose opportunità, ma rischia di farci perdere importanza rispetto a nazioni più capaci di assecondare le necessità delle imprese che lavorano alla *blue economy*. Non possiamo non citare il comparto della pesca, completamente dimenticato, che invece non solo potrebbe rappresentare una leva di occupazione importante, ma che, con i suoi prodotti, può rilanciare un sistema agroalimentare e ittico di alta qualità: basti solo pensare che l'85 per cento del pesce consumato in Italia è di importazione. Per questo e per tanti altri motivi siamo convinti che un Ministero del mare possa mettere insieme tutte quelle competenze che oggi sono sparse in mille uffici diversi - sia che riguardino la cantieristica, le infrastrutture portuali, le regole della pesca o la tutela del mare - ma che, raggruppate sotto un'unica regia, potrebbero dare nuovo slancio all'economia del mare e darci maggiore centralità nel consenso internazionale. La proposta, purtroppo, è stata bocciata: peccato, abbiamo perso un'altra occasione. Noi comunque con la nostra opposizione responsabile e patriottica, che contraddistingue la nostra azione politica sempre per gli interessi degli italiani. In conclusione, signor Presidente, credo di poter dire che che oggi stiamo parlando del riordino dei Ministeri, ma, anche alla luce del dibattito al quale abbiamo assistito questa mattina in Aula, forse la maggioranza dovrebbe concentrarsi sul riordino delle idee, che vediamo alquanto confuse e contraddittorie. *(Applausi)*. Signor Presidente, «il nome racconta la cosa», dicevano gli antichi per cui, quando parliamo di rinomina di nome diverso di un Ministero, dovremmo parlare di un contenuto, non solamente di un'etichetta. Sappiamo che nella fattispecie - ora naturalmente mi concentrerò sul nuovo Ministero della transizione ecologica con questa rinomina, con questa nuova nomina, con questo nuovo nome dovremmo parlare di un nuovo contenuto della cosa cui il nome è dato e assegnato. Storicamente ci apprestiamo ad abbandonare la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» per affrontare un nuovo confine, una nuova possibilità, cioè il Ministero della tanta agognata, quanto detta e annunciata, transizione ecologica. Non siamo la prima Nazione ad aver affrontato un'operazione di questo tipo; sappiamo, per esempio, che altri Paesi europei lo hanno fatto con un certo anticipo, ma noi abbiamo ritenuto che fosse il tempo giusto per affrontare la questione.

che riguarda una nicchia nel contesto delle scelte politiche, istituzionali, sociali e culturali in generale, ma un modo di leggere tutte le politiche. Facciamo attenzione, perché questa è esattamente l'indicazione che viene dall'Unione europea

e quindi col *recovery fund* che non solo è un grande investimento nella logica dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, ma

e se noi mettiamo a repentaglio l'ecosistema del quale siamo parte, mettiamo in discussione il nostro presente e il nostro futuro. Questa è la considerazione culturale di fondo che muove l'operazione dell'Unione europea, il *recovery fund* e dunque la rivisitazione del nome che ridefinisce la cosa.

una visione strategica, una consapevolezza culturale. Qual è la prima grande consapevolezza che ho citato anche prima? Che l'uomo è parte dell'ecosistema e della biodiversità: non esiste una divisione tra l'attività antropica, tra l'essere uomo e il sistema, chiamiamolo creato o come vogliamo, a seconda dei punti di riferimento

perché strutturalmente, ontologicamente l'uomo è persona, dunque è relazione. Questo presupposto culturale mi vede molto favorevole e mi fa dire che la visione della transizione ecologica all'interno di una politica di ecologia integrale non solo è l'unica capace di salvaguardare il pianeta, ma è anche quella necessaria per la crescita economica, per tenere insieme la sostenibilità sociale con quella lavorativa, con quella economica e con quella ambientale. Questa è la visione integrale che parte da una visione culturale per cui persona equivale a relazione, non solo tra le persone, ma con il mondo, con il cosmo ed uso questo termine non a caso, perché è esattamente l'opposto del *caos*, anche nell'antica filosofia. è dunque il luogo in cui l'uomo, costruendo delle relazioni sane, riconosce il valore della natura e costruisce un gioco virtuoso.

l'attività dell'uomo, quando riconosce il valore di una cosa, la rispetta e la riporta a ciò che è in origine, è un'operazione di valorizzazione. Tutela e valorizzazione, quindi, sono esattamente due facce della medesima medaglia.

dopodiché ci sono tutte le ricadute, perché sappiamo che c'è l'attivazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, il cosiddetto CITE, che approva il piano per la transizione ecologica fatto di punti dettagliati, che noi più volte abbiamo posto in quest'Aula e nelle Commissioni: sulla riduzione dei gas climalteranti, la mobilità sostenibile e dolce, il contrasto al dissesto idrogeologico, il contrasto al consumo del suolo, le risorse idriche e le relative infrastrutture, la qualità dell'aria e l'economia circolare. Speriamo vivamente, Presidente, che questo nuovo Ministero definisca, con il cambio di denominazione, un cambio di passo necessario per il futuro nostro e dei nostri figli.

Presidente, signori colleghi, ricorderete che la fenice, il mitico uccello citato anche da Erodoto, rinasceva periodicamente dalle proprie ceneri del tutto rinnovato e più splendido di prima. Vorrei poter usare questa metafora per alludere al neonato Ministero della cultura, ma non posso. Dal 1974 ad oggi, infatti, il Dicastero al quale la Repubblica ha affidato i nostri beni culturali ha cambiato pelle in più occasioni senza mutare la propria essenza. Diversamente, il riordino delle attribuzioni dei Ministeri che oggi affrontiamo sancisce senza dubbio la nascita del Ministero della cultura, ma certifica al contempo l'avvenuto decesso del Ministero dei beni culturali (lo chiamo così per comodità) e la sua è una morte stentata, una morte senza abbandono avrebbe detto il poeta, una morte soprattutto senza speranza di resurrezione. Richiamando il più celebre forse degli elogi funebri, il monologo di Marco Antonio per la morte di Giulio Cesare nell'omonimo dramma shakespeariano, vorrei dire che io vengo a seppellire quel Ministero, non a lodarlo. Franceschini dice che il Ministero dei beni culturali era obsoleto, grave colpa, e che tutti già lo chiamavano Ministero della cultura, quindi non c'è da rammaricarsi del cambio di denominazione e Franceschini è un uomo d'onore. Ma io vengo a parlarvi del Ministero che non c'è più. Dopo l'eccellente lavoro svolto negli anni 1964-1967 dalla Commissione che per beffa del destino si chiamò anch'essa Franceschini, il Ministero voluto da Giovanni Spadolini fu istituito con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. A che scopo un nuovo Ministero? Per attuare l'articolo 9 della Costituzione. Dunque, per garantire la tutela organica di beni di rilevanza assoluta per la Nazione, cioè per il popolo italiano, quali il patrimonio storico artistico e il paesaggio (tutela che è un interesse costituzionale primario) e per gestirli in quell'ottica. Sanità, istruzione e patrimonio culturale sono pilastri costituzionali, ben piantati sulla base solidaristica, irrinunciabili perciò e prioritari.

e, un paio di anni dopo, la legge n. 285 del 1977 garantì carne e sangue alla macchina appena messa in funzione. Le migliaia di giovani assunti in quella stagione sono andati e stanno andando in pensione da circa tre anni, sguarnendo l'organico del dicastero al punto che, teoricamente, esso conta oggi 19.000 unità (da 25.000 che erano prima dei tagli), ma in servizio effettivo ce ne sono appena 12.300, destinati a calare a 10.000 entro il 2025. Con fredda premeditazione non sono state fatte assunzioni per colmare questa emorragia prevedibile e prevista e per trasmettere l'esperienza accumulata. Pensate solo al concorso del 2019 per 1052 assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza (i cosiddetti AFAV), bloccato dopo la prova preselettiva, ufficialmente dalla pandemia, senza che se ne senta più parlare. Meglio per voi ignorare, colleghi, perché che cosa accadrebbe se voi lo sapeste? Dovreste tradire l'uomo d'onore che ha annientato la creatura di Spadolini? Ma torniamo alla storia: con il decreto legislativo n. 368 del 1998 fu istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, che ereditava quanto già spettante al predecessore, con l'aggiunta, però, delle competenze sullo sport e sulla promozione dello spettacolo in ogni sua forma. A fine 2007 fu approvato il nuovo regolamento di riorganizzazione e si intervenne ancora, il 2 luglio 2009, con il DPR n. 91, rafforzando l'azione di tutela e riconoscendo centralità alla salvaguardia del paesaggio. Tutti voi amaste quel Mibac un tempo, colleghi, non senza causa. Quale causa vi impedisce oggi di piangerlo? Il declino è cominciato nel 2013, con il Governo Letta, quando il Mibac rivendica la competenza sul turismo, già della Presidenza del Consiglio. Nasce allora il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo L'onorevole Franceschini, che subentra nel 2014 e che, ad oggi, ha collezionato oltre 1700 giorni da componente dell'Esecutivo, con ben quattro Governi diversi, realizza in un biennio il grosso delle riforme, mandante il presidente del Consiglio Renzi, che stravolgono il dicastero. Si assiste così all'accorpamento degli uffici di tutela, da cui nascono le soprintendenze cosiddette olistiche, esperimento già fallito in Italia negli anni Venti e Trenta, e fallito in Sicilia, dove oggi non sono più garantite le condizioni amministrative per esercitare la tutela, e si assiste al parto, doppiamente mostruoso, dei poli museali e degli istituti con autonomia speciale. È così che la più becera logica spartitoria a fini clientelari si è impadronita della scena, scalzando completamente il merito. Fu allora, colleghi, che il potente cuore si spezzò. Nel 2018, con il Governo Conte 1, si vara il Ministero per i beni e le attività culturali, orfano del turismo associato alle politiche agricole. Già con il Governo Conte 2 e l'inopinato ritorno di Franceschini al Collegio Romano nell'autunno 2019, il giocattolo preferito torna nelle sue mani rapaci per parassitare il Ministero. Io, voi, tutti, cademmo in quel momento. Basti ricordare le decine di milioni di euro sottratti senza esitazioni, lo scorso anno, a quei compiti istituzionali prioritari per finanziare la cosiddetta 18app. Ciò che non produce utili da spartire tra i privati, infatti, non interessa al sinistro della cultura e alla sua corte di rinvenienti, per i quali, come sapete, con il comma 4, soppresso alla Camera, aveva chiesto altri 700.000 euro per il Mic. Ho depositato un emendamento, proprio sulla denominazione del nuovo Ministero, aspetto per nulla marginale. Cultura, infatti, di per sé è un concetto vago e aleatorio, mentre la precedente denominazione conteneva il duplice e distinto riferimento alle funzioni relative: *a)* alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e *b)* alla promozione delle attività culturali, rispettivamente riconducibili ai compiti che i commi 2 e 1 dell'articolo 9 della Costituzione attribuiscono separatamente alla Repubblica. n. 22 del 2021 modificato le precedenti attribuzioni, si deve intendere che la nuova denominazione dovrebbe, logicamente e giuridicamente, ricomprenderle sotto il termine generico di cultura. Sussiste, però, una differenza sostanziale e giuridica fondamentale tra la funzione di tutela dei beni culturali e quella di promozione delle attività culturali, per la diversa natura dei loro oggetti. Mentre il paesaggio e il patrimonio storico e artistico sono compendi di cose (come si esprimeva la legge 1° giugno 1939, n. 1089), ovvero di beni che hanno necessariamente una consistenza materiale individuata di valenza patrimoniale ordinaria, oggetto di tutela, conservazione e restauro (precondizioni della fruizione e valorizzazione della valenza culturale di tali beni), le attività culturali sono comportamenti umani che rilevano per il loro contenuto intellettuale, piuttosto che per gli oggetti materiali che ne sono supporti, strumenti o prodotti, i quali ultimi sono a loro volta oggetto di tutela - e non più di promozione - per i diritti d'autore o quando ne ricorrano le condizioni dell'intervenuto interesse storico quali beni culturali. Un'accezione del termine cultura che dovesse allontanarsi del tutto dalla precedente duplice denominazione forzatamente ricomprendente anche l'effettiva, innominata attribuzione della tutela dei beni culturali e del paesaggio sarebbe pertanto così generica e ampia da creare un illimitato margine di discrezionalità in materia, sovrapponendosi peraltro alle attribuzioni di altri Dicasteri in materia di cultura (alludo a istruzione, università ed esteri). Obliterando tale differenza di funzioni sotto l'eccessivamente generico termine unico di cultura, viene inoltre a crearsi un incongruo disallineamento fra la tutela dei beni culturali e del paesaggio, attribuita al Dicastero dall'omonimo codice e svolta da oltre 640 organi periferici del Ministero e dal 97 per cento del suo personale (mentre la promozione è svolta solo da alcuni uffici centrali), e la sua denominazione. La tutela dei beni culturali come configurata dal codice, pur avendo un presupposto di ricerca e studio e una finalità indiretta di valorizzazione e fruizione culturale, si concretizza in una serie di azioni e procedure giuridico-amministrative relative all'aspetto materiale dei beni, che non possono, per la loro stessa natura, essere considerate mere ed esclusive attività culturali. E non è pensabile, come vorrebbe l'articolo 9 della legge di delegazione europea, estendere oltremodo la definizione di istituti di tutela del patrimonio culturale al fine di favorire l'accesso a quei beni, annacquando il concetto in modo che se tutto è tutela, nulla lo è. L'eliminazione nel Mic di ogni espresso riferimento ai beni culturali costituisce infine un chiaro segnale politico

Occorre pertanto o dare un segnale positivo in senso contrario che dimostri l'intenzione dello Stato di non abbassare la guardia nella tutela dei beni culturali e del paesaggio, restituendo alla denominazione del Dicastero il riferimento espresso ai beni culturali (cioè al patrimonio storico e artistico della Nazione e alla sua tutela che la Costituzione gli attribuisce come compito imprescindibile d'identità e civiltà), oppure che si crei un nuovo Ministero con risorse proprie e un proprio Ministro - vero, non un sicario o un rottamatore - che assolva realmente, con disciplina e onore, a quel compito.

un provvedimento di riordino dei Ministeri (peraltro, mi pare che questa sia la quarta volta che affrontiamo un tema di riordino ministeriale) è sicuramente strategico e molto importante. È questa la fase in cui siamo chiamati a dare l'assetto organizzativo a un pezzo della pubblica amministrazione che, pensando appunto ai due Ministeri più importanti e ai relativi comitati che vengono messi in piedi, dà l'idea

sul nuovo Ministero del turismo, sul Ministero per l'innovazione tecnologica e, di conseguenza, anche sul comitato interministeriale per la transizione digitale.

è componente di diritto del comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; viceversa, di questo comitato non fa parte il Ministero per l'innovazione digitale. Questo un po' preoccupa, perché le due transizioni sono fortemente collegate non nascondo che quadrare il cerchio tra la crescita, l'innovazione digitale e la transizione energetica non sarà così semplice. Comunque sicuramente il Ministero per l'innovazione digitale dovrebbe far parte di diritto di questo comitato. Un'ultima osservazione sul Ministero della della transizione ecologica: si spera che la vera sfida di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e incroci di competenze sia affrontata in maniera effettivamente organica. Qualche dubbio viene, perché il Ministro a capo di questo Ministero, e di conseguenza anche del comitato, potrebbe rischiare di sovrapporsi a una serie di attività, funzioni e obiettivi tipici del nuovo CIPESS (ex CIPE); in questo senso raccomando di evitare le duplicazioni, che sono abbastanza tipiche di questo Paese. Paese. Un altro tema sicuramente molto importante, uno snodo fondamentale, è quello dell'approvazione del Piano per la transizione ecologica, che dovremmo fare entro entro cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge di riordino dei Ministeri. La visione di sistema e soprattutto la forte collaborazione con il Mise

che è molto tipico della cultura italiana. Questi due concetti, quello di *green*,

Arrivo adesso a ciò che a me sta particolarmente a cuore, il nuovo Ministero del turismo. Questo Ministero è stato un po' sballottato, nel senso che non ha mai avuto una sua identità. Ora, io credo che questa identità la debba assumere non solo in relazione alle gravi difficoltà contingenti, che conosciamo tutti e che devono essere affrontate in termini tempestivi, per evitare di distruggere una serie di aziende del settore turistico (mi riferisco a tutto quello che riguarda i prossimi incentivi, i sostegni e quant'altro), ma vorrei che fosse proprio inteso in termini strategici, come vera e propria industria. Qualcuno di voi sicuramente ricorderà che fin dal lontano 2018 io ho detto che il turismo era la più digitale di tutte le industrie. Vent'anni fa, quando Internet era agli albori, nessuno comprese la portata di questo strumento, ma il turismo lo comprese prima di altri settori; questa è l'occasione storica per dare un senso all'industria turistica. Quindi, mi chiedo come questo Ministero, che non è presente nel Comitato interministeriale della transizione digitale, possa svolgere il suo ruolo visto che è la più digitale di tutte le industrie. Sappiamo tutti tutti che anche chi è meno digitale per prenotare un viaggio aereo o una serie di servizi ricorre alle cosiddette piattaforme. Più di una volta ho detto che su questo fronte, cioè su quello che definisco che definisco il digitale immateriale o l'economia digitale, potremmo costruire un pezzo di PIL importante del Paese. Dobbiamo scommettere credendoci perché lì c'è tutto il potenziale inespresso, che anche prima della pandemia non ha dato la sua visibilità in termini di crescita

Titolo V della Costituzione. Mi riferisco all'articolo 117, lettera *r*), della nostra Costituzione, che parla di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. Credo che il dettato di questo articolo debba diventare una parte viva della progettualità digitale della nostra Repubblica in quanto è proprio partendo dal coordinamento digitale che si possono mettere in atto una serie di azioni di sistema. La riorganizzazione ministeriale con la creazione - ripeto - del Ministero dedicato al turismo e di un Ministero dedicato all'innovazione tecnologica deve essere intesa in termini di innovazione organizzativa con una portata di sistema e, quindi, una portata strategica. Dobbiamo declinarlo, in termini operativi e non lasciarlo solo sulla carta. Tale declinazione richiede un atto di coraggio. Penso che l'atto di coraggio sia anche il successivo approfondimento del concetto di *made in Italy*, che ho sempre definito come la sintesi perfetta di bello, buono, ben fatto e bel vivere italiano e, cioè, la sintesi di turismo e di industria creativa italiana. È il modo più concreto per ibridare questi due settori, che poi servono a rilanciare la micro, piccola e media impresa (MPMI) - e non solo la PMI - che rappresenta una parte della spina dorsale produttiva del Paese e che può avvenire attraverso un sistema di valorizzazione digitale che non può scappare dal controllo strategico e che effettivamente può portare nelle «n» nicchie del mondo quanto di meglio l'Italia sa esprimere in termini di eccellenze. Sapete che le eccellenze dell'Italia sono tantissime

dei servizi turistici, ai quali poi andremo a proporre le eccellenze artigianali dell'industria creativa italiana. Mi riferisco alla moda, alla ceramica,

3 punti di PIL. Ricordo ancora una volta a tutti che questo era un comparto che anche prima della pandemia non era sufficientemente valorizzato e promosso nel mondo. È arrivata l'occasione per farlo. Crediamoci e facciamolo.

consentitemi di iniziare con un pensiero per Brumotti, aggredito di nuovo poche ore fa mentre realizzava un servizio per «Striscia la notizia»; al riguardo ci sarebbe tantissimo da dire e per questo preferisco non dire nulla. Mi limito ad esprimergli

del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. Spesso si dice che la forma è sostanza e questo, a mio avviso, dovrebbe già far capire che non si tratta della solita riforma ordinamentale, tra l'altro già realizzata più volte anche in questa legislatura. Ricordo, solo a titolo di esempio, quando furono attribuite le competenze del turismo al Ministero delle politiche agricole e quando, successivamente, nel Governo Conte 2, sempre le competenze del turismo furono restituite al Ministero al Ministero dei beni culturali, scelta che, tra l'altro, io non condividevo e su cui mi ero espresso sempre da questi banchi. In questo caso noi stiamo creando quella che sarà la colonna vertebrale della politica dei prossimi anni, perché questo provvedimento non è fine a se stesso, ma è funzionale alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

in una Nazione piccola (l'Italia ha una superficie di poco più di 300.000 chilometri quadrati), con una popolazione di poco meno di 60 milioni di abitanti. Questo significa che abbiamo una densità abitativa di poco inferiore ai 200 abitanti per chilometro quadrato. Per chi non si dovesse rendere conto di ciò che significa, consideriamo che la Cina ha una densità abitativa di 153 abitanti per chilometro quadrato: l'Italia quindi ha una densità abitativa superiore a quella della Cina. la forte antropizzazione che caratterizza il nostro territorio ci deve far capire che tutto ciò che inciderà sulla politica ambientale dell'attuale Governo, ma anche dei futuri, avrà inevitabilmente ripercussioni dirette sulla vita di tutti noi. Ecco perché, a mio avviso, dovremmo soffermarci sulla portata concreta di ciò che andremo ad Prima di entrare nel dettaglio del contenuto dell'articolo 2, che evidentemente, da membro della Commissione ambiente, mi interessa in maniera particolare, vorrei permettermi una piccola digressione sull'articolo 1, che istituisce il Ministero del turismo. Lo faccio non solo perché è la prima disposizione contenuta nel decreto-legge in esame, ma anche perché, sempre da questi banchi, un anno e mezzo fa, quando si discuteva del trasferimento delle competenze del turismo dal Ministero delle politiche agricole al Ministero dei beni culturali, auspicavo la creazione di un apposito Ministero,

appunto, un apposito Ministero del turismo; quindi, evidentemente, seppur un anno e mezzo dopo, non posso che essere molto soddisfatto di questa scelta. Come dicevo prima, il turismo rappresenta tra il 13 e il 14 per cento del PIL; non è facilissimo fare il calcolo perché poi bisogna considerare anche tutto l'indotto che crea. Ad ogni modo, a prescindere dal fatto che sia il 13, il 14, il 15 o addirittura il 20 per cento, se considerassimo la portata ampia di tutto ciò che è incluso nel mondo turismo, rimane il fatto che tale settore rappresenta un elemento fondamentale per la nostra economia, ancora di più se consideriamo che

che soggetti residenti in altri Paesi portano nel nostro Paese alimentando la nostra economia: 40 miliardi. Se consideriamo che la consistenza totale del *recovery* *fund* è poco più di 200 miliardi, mentre questi 40 miliardi arrivano tutti gli anni, dovremmo capire quanto sia fondamentale per la nostra economia. Oltre alle conseguenze dirette in termini economici, ci sono quelle indirette, perché è evidente che il turismo rappresenta la nostra immagine. Qualche collega prima ha evidenziato

quella privilegiata in assoluto se penso, ad esempio, alla Cina, che equipara la nostra storia, la nostra tradizione, il nostro valore culturale ai loro. Sapendo quanto sono nazionalisti i cinesi, credo che questo dica tutto, che dica tutto, che spieghi in maniera esaustiva quanto l'immagine dell'Italia all'estero sia un valore enorme, di cui forse nemmeno noi ci rendiamo sempre conto. Ecco perché valorizzare il turismo significa valorizzare la nostra immagine e consentire la realizzazione appieno di quel progetto di *made in Italy* che dovrebbe essere finalizzato non solo alla tutela dei nostri prodotti, ma anche alla loro promozione all'estero. L'ultima considerazione per cui, a mio avviso, il turismo è fondamentale - consentitemelo con una una nota di evidente orgoglio - è perché sono marchigiano: vengo da quella Regione che la rivista «Lonely Planet» ha indicato come la seconda più bella al mondo. Quindi, tutte queste motivazioni inevitabilmente mi portano a pensare che la realizzazione del Ministero del turismo sia stata una scelta utile e opportuna, forse un po' tardiva, ma, come si dice sempre, meglio tardi che mai.

l'impedimento per la prosecuzione dell'attività. Non possiamo, quindi, limitarci esclusivamente a mantenere la politica dei piccoli ristori che c'è stata fino ad ora, ma dobbiamo fare tutto quanto necessario affinché questo settore possa ripartire. Penso, ad esempio, alla ristorazione.

che quella rappresenti la soluzione ideale - e, oltre ad aver mangiato il panino in quella maniera, evidenzio che avevamo accanto forse una quindicina di altre persone che erano state costrette a fare la stessa cosa. Quindi, nell'ottica di ripartenza di questo settore, teniamo anche in considerazione le proposte di buonsenso che vengono dalla Lega per le riaperture e per la gestione dei prossimi mesi, che saranno fondamentali. *(Applausi)*. Se parliamo di turismo, un mese non vale l'altro: agosto non è uguale a marzo o a febbraio. L'indotto, le attività, il fatturato, l'economia che abbiamo perso nelle nostre montagne con la chiusura degli impianti sciistici non li recupereremo più per quest'anno. dobbiamo capire che serve ed è indispensabile fare qualcosa adesso... Arrivo subito alle competenze attribuite al Ministero per la transizione ecologica. Tale Ministero ha competenze vecchie, che eredita dal vecchio Ministero dell'ambiente, ma anche competenze nuove. Evidenzio che quando si parla di transizione ecologica, si deve tener conto che si corre il rischio enorme di ideologizzare delle scelte e la politica di questo Ministero, senza rendersi conto

significa avere, come conseguenza immediata, il fatto che chi pensava di cambiare una macchina vecchia per una nuova non lo fa, in attesa di sapere quale sarà la politica del Governo al riguardo. Pertanto, l'intenzione e la volontà sarebbero quelle di migliorare quelle che sono le emissioni in atmosfera di gas inquinanti, ma in realtà il risultato ottenuto è che tenendo le macchine vecchie, non si ottiene più il risultato voluto.

che queste decisioni, avendo conseguenze dirette sulla vita di tutti noi, dovranno essere ben ponderate, ma soprattutto concrete. *(Applausi)*.

dal mese di febbraio l'Italia è il terzo Paese al mondo ad essere dotato di un Ministero per la transizione ecologica. Questo super Ministero unisce le competenze del Ministero dell'ambiente a quelle del Ministero dello sviluppo economico in materia di energia e nasce insieme ad un organismo estremamente importante collocato all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri, che prende il nome di Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Questo Comitato, presieduto dal Capo del Governo, con il Ministro per la transizione ecologica come vicepresidente, ha il compito di assicurare il coordinamento di tutte le politiche nazionali per la transizione ecologica, come la riduzione delle emissioni di gas climalteranti, la mobilità sostenibile, il contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo, l'adattamento ai cambiamenti climatici, le risorse idriche, la qualità dell'aria, l'economia circolare e i sussidi ambientali. La ragione della presenza del MoVimento 5 Stelle nel Governo è esattamente questa: la nascita del Ministero per la transizione ecologica e del Comitato interministeriale per la transizione ecologica. La transizione ecologica e solidale è stata difatti la condizione non negoziabile che abbiamo posto al presidente Draghi per partecipare al suo Governo di unità nazionale. Oggi ci troviamo infatti a vivere un momento storico unico e irripetibile. Cominciamo con fatica ad intravedere la possibilità di uscire dalla crisi di sistema provocata dal Covid. La crisi ha causato danni enormi sul piano sanitario, sociale ed economico, che il Paese sta ancora subendo, ma siamo tutti fiduciosi nel fatto che tra qualche tempo ci si possa concentrare sulla ripresa. Questo, come dicevo, è un momento storico eccezionale; abbiamo un Paese da ricostruire, abbiamo a disposizione un'ingente quantità di denaro, delle linee guida europee molto precise riguardo l'utilizzo dei soldi per la sostenibilità ambientale e un Governo di unità nazionale presieduto da un Presidente del Consiglio forte sul piano internazionale. Ci sono quindi tutte le condizioni per fare quel cambio di passo verso la transizione ecologica che il MoVimento 5 Stelle chiede da sempre e che dovrà necessariamente coinvolgere tutte le forze politiche. Tutte dovranno iniziare a pensare al futuro del nostro Paese da qui al 2050. Il Ministero della transizione ecologica e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica avranno il compito di coordinare l'azione dell'intero Governo per affrontare in modo trasversale le tre grandi crisi che stiamo vivendo: la crisi sociale, la crisi ecologica e la crisi economica. Partiamo dalla crisi sociale. La transizione non sarà solo ecologica: sarà una transizione ecologica e solidale. Se vogliamo che tutti i cittadini vi partecipino attivamente, dobbiamo sollevarli dalla precarietà economica e dalla paura del domani, riducendo le disuguaglianze. La transizione è di tutti e per tutti, oppure non sarà per nessuno. Per quanto riguarda la crisi ecologica, i problemi della sostenibilità sono conosciuti da almeno settant'anni, ma finora abbiamo fatto pochissimo. Siamo abituati a rincorrere e tamponare le emergenze del presente, rinviando al futuro le soluzioni, senza intervenire sulle cause e senza preoccuparci delle conseguenze a lungo termine. Avviare la transizione ecologica e solidale richiede alla politica un cambio di prospettiva: agire nel presente, certo, ma per costruire l'Italia del 2050. È un impegno che spetta non solo al MoVimento, ma a tutte le forze politiche. L'urgenza del 2021 e la previdenza per il 2050 devono combinarsi, non ostacolarsi. Nella transizione il tema dell'energia è importante, ma la soluzione non è semplicemente passare dall'energia fossile a quella rinnovabile; occorre un cambiamento molto più ampio che coinvolga abitudini, stili di vita, mentalità e obiettivi. Finora abbiamo orientato tutti i nostri sforzi per ottenere più produzione, più lavoro, più guadagni, più cose. Con la transizione riconosceremo il valore delle persone, della qualità del lavoro, del tempo, delle relazioni e della vita. Useremo l'intelligenza per vivere con più soddisfazione ma con meno energia, meno materiali, meno lavoro a pari livello di benessere. Lo *slogan* deve essere: meno potenza, più intelligenza.

Mette a rischio l'economia, la crescita, la finanza, causa disoccupazione, povertà e migrazioni. Tutto questo è un costo economico altissimo, un costo enorme che aumenta sempre di più per effetto del nostro ritardo. Sono cinquant'anni che continuiamo a rinviare il cambiamento. Anche la transizione ecologica avrà un costo, è vero, ma sarà comunque molto inferiore al costo di non farla. Nel 2006 l'economista britannico Stern calcolò che agire sul clima subito sarebbe costato dieci volte meno che non farlo; oggi, nel 2021, dopo quindici anni, il costo del non agire è quasi raddoppiato. Al di là delle diverse sensibilità ambientali, è evidente che le motivazioni economiche per attuare la transizione ecologica sono fortissime e chiamano in causa tutte le forze politiche, tutte le forze politiche, che devono avere la lungimiranza di guardare all'Italia del 2050. L'Italia è tra i primi Paesi al mondo a impegnarsi in questa sfida. Qualcuno non si convincerà facilmente (è normale), anni Settanta nessuno capiva il senso del Ministero dell'ambiente creato in Nuova Zelanda; poi col tempo però tutti i Paesi ne hanno istituito uno. La direzione, quindi, è chiara: nei prossimi anni la transizione ecologica arriverà al centro dell'agenda politica di moltissimi Paesi. Sulla transizione ecologica non ci si può dividere tra destra e sinistra, non ci sono ideologie che tengano: è la realtà a imporci un cambiamento necessario e urgente. Tutte le forze politiche da qui al 2050 sono chiamate a raccogliere la sfida, a dare il loro contributo con il massimo impegno. La transizione ecologica non è una bandiera del MoVimento 5 Stelle, deve essere una bandiera di tutti e per tutti

ma che vada solo aggiunto il nuovo scopo, la nuova missione che il Ministero si dà. Quindi esso dovrebbe denominarsi, più propriamente, Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della transizione ecologica "Mattme". è infatti un termine che, non a caso, è usato molte volte nella nostra Costituzione, perché sta ad indicare un preciso obbligo, a difesa di un preciso diritto

È vero, la transizione ecologica oggi è una priorità e riguarda tante delle azioni inerenti alla tutela, perché risponde alla necessità non più derogabile di ridurre quell'impronta ecologica che grava sul nostro pianeta a causa dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. La transizione, tuttavia, denota solo una missione, un'esigenza, uno scopo che il Ministero si propone di mettere in atto per transitare, ossia per

da apposito Ministero, dal Mise, per esempio. Questi sono gli stessi ragionamenti alla base della proposta al punto 11), per cui si chiede che il Ministero dell'istruzione torni a chiamarsi Ministero della pubblica istruzione,

nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (che sappiamo tutti che compiti svolge, attinenti la politica per l'informazione e la sicurezza), chiedo se possa essere inserito anche il Ministero il Ministero dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, visto che c'è affinità di contenuti.

Noi riteniamo opportuno che di questo Comitato faccia parte anche il Ministro del turismo, alla luce del fatto che il turismo è un'attività antropica che, oggi più che mai,

«a provvedere ad una puntuale ricognizione dei compiti attribuiti ai commissari governativi già in essere, valutando l'eventuale razionalizzazione, con l'obiettivo di rendere più agevole ed efficace la programmazione e la gestione dell'attività».

e territoriale, garantendo che le risorse economiche stanziate dallo Stato e dall'Unione europea per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecosostenibile del territorio vengano impiegate in base ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, semplicità e trasparenza;

che non è mai stata risolta da nessun Governo ad oggi. È stato trasformato in ordine del giorno, che la Commissione ha accolto e che ringrazio per il lavoro svolto.

approfondendo il contenuto degli stessi, si valuta come servano a ridefinire il profilo dell'azione di Governo, come in questo caso. Sono quindi provvedimenti che hanno l'obiettivo di ricostituire la struttura del Governo, secondo precise scelte politiche e secondo priorità che il Governo intende quindi una rivisitazione legittima dell'assetto del Governo, corrispondente sicuramente ai bisogni che oggi si avvertono per quanto riguarda le risposte che occorre dare alla società a fronte delle richieste avanzate, per soddisfare quei bisogni

dà, infatti, una struttura al Governo, ridefinendo gli assetti ministeriali sulla base di alcuni importanti principi, soprattutto dando alla struttura dei Ministeri una connotazione politica attraverso le parole chiave che vengono inserite nelle diciture che li identificano. Transizione ecologica, mobilità sostenibile, innovazione tecnologica, turismo, sviluppo economico: sono questi i temi che emergono

delle quali hanno su questo una predisposizione e un impegno politico maggiore di altre. Ad ogni modo tutto il Parlamento è sicuramente interessato e impegnato sul tema della transizione ecologica. In questo senso, anche Italia Viva ha svolto un proprio lavoro di approfondimento e di condivisione, attraverso un emendamento che è stato approvato alla Camera, che ha previsto la possibilità di far partecipare il Ministro della transizione ecologica al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, proprio partendo dalla

la struttura del Governo per dare risposte in una fase politica e sociale complicata, quella *post* pandemica, gli effetti della pandemia non sono sicuramente da considerare esauriti, ma sono ancora importanti. È chiaro che dobbiamo dare delle risposte perché serve una pubblica amministrazione preparata, organizzata, all'altezza della sfida

aperto una conflittualità tra Governo e Parlamento; ricordiamo tutti la fase dei famosi DPCM, che poneva all'attenzione un contrasto tra il potere decisionale del Governo e la capacità di incidenza Dobbiamo superare quella contrapposizione; ci deve essere una dialettica costruttiva. Chiaramente, rafforzando il Governo, si deve rafforzare anche la capacità

come avverrà nelle prossime settimane con il provvedimento che sancisce le prime riaperture a partire dal 26 aprile, si è scelta una strategia di maggiore coinvolgimento del Parlamento, che dovrà convertire

consentirà di dare risposte efficaci e tempestive soprattutto alle imprese e alle famiglie, che sono i soggetti che stanno pagando più duramente in questa fase complicata Dobbiamo dare risposte, quindi, per combattere il disagio e per accompagnare la nuova stagione di riapertura del Paese, che gran parte dello stesso si aspetta per tornare alla vita reale e ridare slancio all'economia.

combattere il virus e dare un segnale chiaro di ripartenza delle attività e della vita, intendiamo esprimere un voto favorevole a questo provvedimento. Siamo convinti che di un'ulteriore spinta affinché le politiche del Governo e il rapporto con il Parlamento consentano di ridare slancio al Paese e una prospettiva nuova dopo questa fase complicata di gestione degli effetti della pandemia.

come Fratelli d'Italia ci dispiace dover esprimere un voto contrario su questo provvedimento che riguarda un aspetto istituzionale della vita del Governo e del Parlamento, ovvero il riordino dei Ministeri. Ci dispiace doverlo fare perché, nel farlo, dobbiamo evidenziare che alla base di questo riordino non vi è nulla di quello che avrebbe dovuto determinarlo.

e rende più difficile il compito del Parlamento nel confrontarsi con il Governo nell'esercizio dei suoi poteri. Lo facciamo e lo diciamo ben sapendo che oggi - mi rivolgo soprattutto alla sinistra che ha ereditato dalla Democrazia Cristiana la presunzione di essere il partito delle istituzioni, che una volta era rappresentato, appunto, dalla Democrazia Cristiana, alla sinistra, erede in parte di quella tradizione, che ha avuto la presunzione di di interpretare il senso dello Stato e delle istituzioni a prescindere e che invece non fa più questo da tempo e non lo fa certo con questo provvedimento - è proprio la destra italiana a dover assumere su di sé la responsabilità di garantire la legalità democratica, di garantire il buon funzionamento del Parlamento, dei suoi organi esecutivi e dei suoi comitati di garanzia. È proprio la destra italiana che deve farsi carico, nell'assenza di un partito della maggioranza che lo faccia pienamente, di bilanciare l'efficacia dell'Esecutivo con i compiti del Parlamento.

ad inizio legislatura. Ciò è avvenuto con il Governo Berlusconi del 2001, che ha applicato, per la prima volta in modo compiuto, la riforma Bassanini con l'accorpamento dei Ministeri e lo ha fatto anche se quella riforma era stata elaborata dalla sinistra. Chi ha senso dello Stato, infatti, non cambia lo Stato con il cambiare del Governo. *(Applausi)*. Il Governo Berlusconi applica la riforma Bassanini. Io fui delegato al commercio con l'estero, che fu accorpato, per effetto di quella riforma, al Ministero dello sviluppo economico, allora Ministero delle attività produttive.

che quando si accorpa o si scorpora un Ministero, quando si cambiano le funzioni di un dipartimento, per realizzare il provvedimento ci vogliono poi Ci vogliono anni per trasferire il personale, le competenze e per poterle esercitare. Ci vogliono anni. Per tale ragione prima si operava ad inizio legislatura. Così accadde nel 2001, così accade con il Governo Prodi nel 2008. La sinistra, La sinistra, che aveva realizzato la riforma Bassanini accorpando i Ministeri, tornata al Governo con Prodi, scorpora i Ministeri; il commercio internazionale torna ad essere un Ministero e così anche altri. perde, senza accorgersene, l'anima istituzionale, sacrificandola agli interessi politici. Comunque lo fa all'inizio della legislatura e la collega Bonino diventa Ministro per il commercio internazionale, a sua volta scorporato e, allo stesso tempo, Ministro per le politiche europee, due deleghe in una; legittimo, ma siamo all'inizio della legislatura. Così accade anche quando Berlusconi torna al governo nel 2008. All'inizio della legislatura riaccorpa i Ministeri, seguendo l'architettura dello Stato di Bassanini, che la sinistra ha ideato e non realizzato. Vi rendete conto di quello che state facendo? Come vi siete trasformati nell'anima, perdendo quella funzione di legalità democratica e istituzionale? Comunque viene fatto ad inizio legislatura. Noi ci assumiamo la responsabilità di seguire la riforma dei Ministeri indicata dalla riforma Bassanini, e accorpiamo i Ministeri che voi avete scorporato. Personalmente torno a fare il Vice Ministro. Veniamo però alle legislature successive. A un certo punto,

due modifiche di poco conto perché ancora comunque permane un senso della cultura dello Stato: in Letta, certamente, e dopo in Renzi. Veniamo a questa legislatura.

ma non basta però un anno per applicare le disposizioni che riformate: è un gioco dell'oca! Vi siete appropriati delle istituzioni e le asservite agli interessi politici, talvolta agli interessi personali Non vi rendete conto di quello che state facendo al senso dello Stato che dovete trasmettere cittadini. L'esempio è eclatante con il Ministero del turismo: nel primo Governo di questa legislatura

Non ci siamo! Non potete utilizzare le istituzioni a vostro piacimento! Non ci siamo, non potete asservire lo Stato alle logiche degli interessi politici o personali.

Così non va, non può andare anche laddove c'era una visione giusta, come sul digitale. Però non basta cambiare nome al Ministero dell'innovazione per farne il traino della nuova economia del Paese,

ma la destra italiana sa che deve agire in questo Parlamento e in questo tempo per salvaguardare le istituzioni, il bilanciamento dei Poteri e le regole democratiche che purtroppo, con la dimostrazione odierna, calpestate. È iscritta a parlare la senatrice Pavanelli. Ne ha facoltà. Signor Presidente, personalmente mi limiterò a toccare solo alcuni temi che ho sentito durante questo dibattito, perché credo che il decreto-legge in esame sollevi dei punti a cui è giusto dare una risposta ed è giusto farlo anche quando - e credo sia questo il caso provvedimento arriva con un sostegno parlamentare e nella maggioranza molto ampio, a cui il Partito Democratico ha dato un contributo che oggi ribadiamo con convinzione.

di modellare l'organizzazione dell'Esecutivo sulla base del suo piano di programma, quel programma che ha ricevuto la fiducia del Parlamento. Questo chiaramente non vuol dire fare e disfare tutto ogni volta e, d'altra parte, non sarebbe questo il caso. Ma è evidente che ciascun Governo ha la comprensibile esigenza di darsi una struttura ministeriale e amministrativa coerente col proprio indirizzo politico, sempre muovendosi all'interno della cornice stabilita dalla legge n. 400 del 1988, che è e resta il faro ordinamentale di questo campo. È chiaro però che un progetto politico deve trovare supporto in una struttura e per questo la struttura deve poter avere una sua determinata flessibilità. C'è poi una seconda questione, alla quale tengo di più, in questa fase così particolare come quella che stiamo attraversando. Abbiamo concluso poche settimane fa un dibattito fondamentale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui abbiamo fornito, ciascuno secondo le proprie legittime proposte, proposte, suggerimenti per utilizzare al meglio la grande mole di risorse che potremmo avere a disposizione grazie al Piano europeo di sostegno. Ecco, in quella discussione, tutti, in maniera condivisa, abbiamo riconosciuto che transizione digitale e transizione ecologica sono due assi strategici su cui si costruirà il futuro del nostro Paese. Io aggiungo che, se questo è vero, non è però scontato che quelle stesse trasformazioni siano di per sé eque, inclusive e democratiche. I cambiamenti che abbiamo all'orizzonte, a partire - per esempio - dalle misure contro il cambiamento climatico, produrranno effetti sui cittadini e sulle famiglie; effetti che hanno bisogno di essere governati, altrimenti il rischio è che impattino in maniera profondamente disuguale e iniqua sui cittadini. Ma se è vero quello su cui tutti abbiamo concordato nel dibattito sulla relazione del PNRR, allora oggi con questo decreto noi possiamo - io dico dobbiamo - essere conseguenti e coerenti, poiché quelle erano scelte di indirizzo politico; oggi invece diventano i palinsesti concreti e materiali per mettere in campo quella precisazione di Governo. Le due scelte fondamentali di questo decreto - da un lato, quindi, Ministero per la transizione ecologica e, dall'altro, Ministero per la transizione digitale - credo siano esattamente la coerente e logica prosecuzione di quelle prospettive su cui ci sono stati un dibattito e una condivisione prima nelle Commissioni e poi qui in Aula. Aggiungo poi un elemento che mi pare degno di nota: c'è stato chi ha sollevato qualche perplessità sul fatto che dietro il nuovo assetto del Ministero per la transizione ecologica ci sia un impianto ideologico che metterebbe in contrasto tutela dell'ambiente e sviluppo economico del Paese. Paese. Su questo tema dovremmo tutti ricordarci che questioni simili vennero sollevate in maniera trasversale quando fu istituito nel 1986 il Ministero dell'ambiente. E abbiamo visto negli anni successivi che quei rischi non solo non c'erano, ma erano addirittura esagerati, e l'esperienza ha dimostrato che non è stato affatto un ostacolo il Ministero, così inteso, allo sviluppo economico e industriale del Paese, ma è stato una sua preziosa risorsa. Aggiungerei che si tratta anche di una garanzia, soprattutto dal punto di vista dei rapporti con le Regioni, perché la presenza di un Ministero dell'ambiente al tavolo del Consiglio dei ministri ha portato a impegnative leggi regionali, della Costituzione, andavano contro una moderna tutela dell'ambiente. Se guardiamo all'oggi c'è ancora di più: le scelte compiute dal decreto in esame in fatto di competenze e di funzioni di questo Ministero, a partire naturalmente dall'ambito delle politiche energetiche e minerarie, sono la premessa affinché esso diventi un punto di riferimento per orientare tutte le politiche verso un obiettivo di sostenibilità che deve essere nazionale e che si muove in un contesto globale. In questo non c'è alcuna matrice ideologica, non c'è alcuna contropartita offerta per tenere insieme la maggioranza, cose che pure ho sentito. C'è invece la volontà concreta di raggiungere un obiettivo, da cui passerà verosimilmente la modernizzazione del nostro Paese. Lo stesso direi che vale per il Ministero per la transizione digitale, che avrà un ruolo di coordinamento importante su azioni di riforma che - come ben sappiamo - dovranno necessariamente essere trasversali. Aggiungerei che anche la scelta di dare una competenza mirata e autonoma sul turismo, su cui da tempo si discuteva e che dopo quest'anno di pandemia diventa inevitabile, non è soltanto una scelta simbolica, ma è anche lo sbocco quasi naturale di un'esigenza reale e assolutamente non strumentale. Un ultimo punto che è stato sollevato in discussione e che è effettivamente delicato riguarda le procedure adottate per la riorganizzazione dei Ministeri. Sappiamo che la riorganizzazione interna è demandata alla procedura prevista dalla legge n. 400 del 1998, che è effettivamente articolata in molti passaggi. La prova ne è il fatto che dal 2012 si adotta una procedura semplificata, attraverso decreti del Presidente del Consiglio in deroga e che ora sono riprodotti anche dal decreto in esame. Tutti vedono i vantaggi di questo percorso, perché evita le complicazioni dell'articolo 17 della citata legge, dà maggiore flessibilità all'organizzazione dei Ministeri, in questo modo viene saltato il parere delle Commissioni, che invece è previsto dal procedimento ordinario. Probabilmente per il decreto-legge in esame non c'erano altre strade; ma, se da anni viene usata la soluzione in deroga, è il segno di una funzione reale che esiste. Per il futuro qualcosa di diverso si può cercare, per tenere in equilibrio sia esigenze di semplificazione e flessibilità, sia la partecipazione del Parlamento, perché è nel coinvolgimento reciproco di Parlamento e Governo che sta in piedi il nostro sistema. In conclusione, ho fatto riferimento ai tre cambiamenti che sono l'asse portante di questo provvedimento, ma sono soprattutto una scelta coerente e giusta, oltre che pienamente legittima. È questo il motivo per cui voteremo a favore però, c'è anche una sfida che tutti i soggetti investiti dovranno saper cogliere; una sfida culturale che investe la politica, ma che vede coinvolti anche i livelli competenti delle amministrazioni ministeriali. Il senso di costituire livelli di decisione trasversali tra competenze ministeriali diverse regge, se poi questi comitati funzionano e hanno un'efficacia reale. Se invece il centro decisionale si sposta all'esterno, da un'altra parte, la loro funzione resta soltanto nominale e credo non sarebbe un bene. In questa direzione è un buon segnale, pur soltanto iniziale, il coinvolgimento del Parlamento, con il parere delle Commissioni di merito, nel piano per la transizione ecologica proposto dal nuovo Comitato interministeriale per la transizione energetica. È questa la strada che dobbiamo perseguire, affinché quello che oggi ci apprestiamo a modificare nella struttura dei Ministeri si affermi anche nella qualità delle politiche, come un vero elemento di novità, concreta e duratura nel tempo. Per queste ragioni, esprimo il primo il voto favorevole del Partito Democratico.

per ricevere il voto di fiducia, ma dalle indicazioni e dal profilo programmatico discendono giustamente delle conseguenze dal punto di vista della trasposizione operativa. Questo è il punto

la transizione comporta anche la transizione dei modelli produttivi, con indicazioni chiare e la costruzione intorno a questo punto di una politica industriale.

cancellare quelle che sono state le competenze storiche e primarie del Ministero dell'ambiente, che nel tempo si era trasformato in Ministero della tutela del territorio - sappiamo cosa significa tutela del territorio, cosa significa governare e

un Paese che ha ancora una ricchezza, purtroppo messa a repentaglio giorno dopo giorno, ma sicuramente di primato a livello europeo.

con personale preso da una parte e dall'altra. Oggi non basta soltanto creare un grande Ministero e cambiargli nome, ma bisogna anche dargli e mettere in campo i mezzi, gli strumenti, le qualifiche e il personale

interministeriale per la transizione digitale è fondamentale, e ci siamo accorti in questa pandemia di quanto tempo perso abbiamo dovuto recuperare.

del turismo è stata ceduta al Ministero dei beni culturali. Ora lo scorporiamo di nuovo dal Ministero dei beni culturali. il modo in cui affrontiamo la questione del turismo, che tra l'altro oggi è un'emergenza vera e propria, perché si tratta di ricostruire completamente le politiche del turismo, che è un settore che è stato quasi distrutto dalla dalla pandemia e per fare ciò serve avere le idee chiare e sapere che tipo di rilancio si può fare. Devo constatare che, nel passaggio da un Ministero all'altro, forse si sarà consumata tanta carta a forza di cambiare intestazione, ma certamente non ci siamo soffermati su delle scelte nell'ambito delle politiche industriali.

ci arriva dalla Camera questo provvedimento che mi piace pensare sia stato il frutto non di una becera spartizione all'interno di una maggioranza, peraltro neanche omogenea, ma della necessità di razionalizzare l'organizzazione di alcuni Ministeri in vista e in prospettiva dell'utilizzo degli oltre 200 miliardi di euro che di qui a qualche mese - ci auguriamo il più presto possibile - arriveranno nel nostro Paese. credere - è stata un'iniziativa idonea e necessaria, e lo valuteremo nel tempo e lo valuteremo a consuntivo, dopo che sarà portato

se si parla soltanto di cambiamento del nome, evidentemente non abbiamo colto nel segno Credo vi sia una filosofia completamente diversa nel Ministero della transazione ecologica, che ha grandissima importanza. E ritengo che una delle finalità delle risorse che arriveranno dall'Europa sia proprio la transizione

di fare formazione alle imprese, di dare sostegno alle imprese perché si abbia un circuito virtuoso nel quale poter inserire anche

ma avrebbero poco senso se la finalità del nuovo Ministero non fosse anche quella di venire incontro alle esigenze del mondo produttivo, ma fosse soltanto di sanzionare e di porgersi in maniera alternativa allo sviluppo industriale Lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo con la tragedia dell'Ilva - constatando come il nostro Paese sia arretrato nella produzione dell'acciaio - e lo abbiamo visto anni fa con la chimica fine che abbiamo trasferito a gruppi stranieri, venuti con la scusa di salvare l'occupazione ma interessati soltanto ad acquisire le quote di mercato, che ci hanno lasciato gli impianti inquinanti e anche la disperazione della disoccupazione. che questo Ministero abbia un ruolo nevralgico nel PNRR del nostro Paese. Un'altra novità, che poi è un ritorno al passato, è la costituzione del Ministero del turismo. Siamo stati facili profeti quando, due anni fa,

un ganglio fondamentale dell'economia nel nostro Paese e dobbiamo concorrere e competere con Paesi che, soltanto pochi anni fa, ci guardavano da lontano e che oggi siamo costretti a inseguire: parlo della Grecia, parlo della Spagna, ma anche della Croazia. Quindi, il Ministero del turismo è un altro elemento fondamentale ed è stato giusto - dal mio punto di vista - dargli la dignità di un Ministero proprio per il fatto di essere un elemento cruciale nella nostra economia. Anche in un momento di pandemia, che ci auguriamo di metterci alle spalle quanto prima, è determinante e fondamentale l'attività del Ministero del turismo, soprattutto in vista delle prossime riaperture; riaperture

Una modifica introdotta alla Camera introduce il Ministero della transizione ecologica nel Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, organo di raccordo politico strategico sul tema della sicurezza nazionale. Questa è ancora di più la prova di quanto sia cruciale e nevralgico detto Ministero, come è cruciale nascita di alcuni comitati interministeriali che rimangono nella responsabilità e nella direzione della Presidente del Consiglio. Quello della transizione ecologica e digitale è un altro appuntamento a cui il nostro Paese non può e non deve mancare. mancare. Una digitalizzazione della pubblica amministrazione rappresenta una spinta enorme all'economia del nostro Paese,

Altro è stato detto e non ritengo che sia opportuno e necessario ripeterci. Voglio soltanto, avviandomi alla conclusione, parlare del MIMS, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Anche in approfittiamo delle risorse europee per cercare di diminuire e azzerare il *gap* esistente tra il Nord e il Sud. Esistono territori

Quindi, quando si parla di mobilità sostenibile, si deve intervenire e operare perché tutto il territorio nazionale abbia le stesse opportunità. Si parla tanto della questione meridionale; si parla tanto del fatto di essere vicini al Mezzogiorno. Il Mezzogiorno non vuole prebende; il Mezzogiorno non vuole assistenza; il Mezzogiorno vuole riconoscimento della propria dignità e vuole le pari opportunità. Vuole avere le stesse opportunità che si hanno nelle altre Regioni del nostro Paese. Io credo che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile sia assolutamente essenziale per questo tipo di attività. Allora, pur avendo voluto apportare alcune modifiche al provvedimento in esame (modifiche più di *drafting* che di sostanza), ci rendiamo conto che i tempi nei quali è arrivato al Senato della Repubblica impediscono

riorganizzare i Ministeri è non soltanto un esercizio di diritto amministrativo, ma anche un'attività strettamente funzionale all'azione politica che un Governo intende esprimere. In quest'occasione, tra l'altro, la riorganizzazione dei Ministeri è particolarmente importante perché l'attuale Governo nasce con lo scopo principale di gestire una gravissima crisi determinata da una delle 10 più gravi pandemie che abbiano mai colpito l'umanità. Sono sotto i nostri occhi le conseguenze economiche di questa pandemia. Sappiamo, dunque, che adesso a noi tocca il compito di guidare la ricostruzione economica dell'Italia, oltreché - ma è superfluo dirlo - guidare il Paese verso il recupero della serenità e del buono stato di salute. Non dimentichiamo, poi, che bisogna gestire i fondi del *recovery plan*.

penso al Ministero del turismo. Il turismo è il settore che maggiormente ha subito le conseguenze della pandemia. Sappiamo che il turismo determina una quota molto importante del PIL del Paese e che senza di esso l'economia italiana non può ripartire. Bene, dunque, dar vita in modo autonomo a un Ministero del turismo che sia in grado di promuovere specifici interventi per il settore. Si tratta di un segnale chiaro che questo Governo lancia al Paese. Era il momento giusto per far confluire tutte le funzioni statali in materia di turismo sotto un unico Ministero, in modo da consentire di mettere in campo strategie oltre un'ottica emergenziale. Il turismo italiano viene perciò slegato

all'azione politica di concentrarsi sul rilancio del turismo come movimentazione di denaro. Un altro aspetto sostanziale riguarda la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero

L'intenzione dichiarata è di voler lavorare su politiche più sostenibili. Come Gruppo riteniamo sicuramente importanti la valorizzazione e la protezione delle risorse naturali e come maggioranza vogliamo lavorare per questo obiettivo. Confidiamo nella ricerca di un giusto equilibrio - questo è un passaggio molto importante - tra la tutela dell'ambiente e le politiche di sostegno ai settori produttivi. Attenzione: è importante che questo Ministero persegua politiche *green* intelligenti, perché non sempre ciò che appare sotto l'insegna dell'ecologia e della tutela dell'ambiente è davvero tale. In alcuni casi una politica *green* può infatti semplicemente portare a nascondere sotto al tappeto la polvere e l'immondizia. *(Applausi)*. all'uso dell'elettrico: ormai c'è una tendenza mondiale alla trasformazione del parco circolante in parco a trazione elettrica, ma gli studi più avveduti ci lanciano un allarme, segnalando che la transizione irragionevole verso l'elettrico rischia di portare a un'altra forma di inquinamento. Pensiamo allo smaltimento delle batterie e anche ai rischi legati all'approvvigionamento delle materie prime. Vorrà dire che sposteremo la nostra attenzione verso altri Paesi, dove è possibile trovare i materiali necessari alle produzioni di queste batterie. Quindi attenzione, perché questa sfida *green*, se è vero - come è vero - che è anche un'occasione di crescita, non deve trasformarsi in un boomerang per gli interessi di questo Paese. Ci vuole studio; ci vogliono gli investimenti nel campo della ricerca e della tecnologia affinché il Paese sia in grado di compiere scelte ecologiche ragionevoli e sostenibili. Lo stesso monito, fatti fatti gli opportuni adeguamenti, possiamo utilizzarle per la transizione digitale: sappiamo che è stato istituito questo importante Ministero. Intenet, ha sicuramente cambiato la storia dell'umanità e ancora non ne vediamo compiutamente gli effetti, perché siamo osservatori troppo coinvolti per poter comprendere l'importanza di quello che sta accadendo. All'indomani della scoperta della stampa ad opera di Gutenberg - stiamo parlando della prima metà del Quattrocento - ancora l'umanità non si era resa conto di quello che stava per accadere; anni dopo è iniziata la Rivoluzione industriale. Con Internet tutto sarà più rapido, ma anche in questo caso dobbiamo capire che il digitale, le informazioni, i dati, la gestione dei dati sono nozioni che richiedono un nuovo modo di pensare. Guai se pensiamo di utilizzare Internet secondo i nostri vecchi schemi; che il digitale non sia uno strumento della pubblica amministrazione per aumentare la complessità delle procedure a danno dei cittadini. Le norme dovranno essere scritte in funzione della maggiore velocità di accesso ai dati tramite Internet. La Lega guarda con favore all'istituzione di questi Ministeri, ma lancia un monito: questi strumenti politici e amministrativi siano utilizzati con intelligenza, con cultura e competenza. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del partito cui appartengo, cioè la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

che ridefinisce le funzioni dicasteriali in materia di energia, turismo e di innovazione digitale e provvede a rinominare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Per il Mite, il Ministero della transizione ecologica, si è dato vita a una struttura che è in grado di utilizzare quel poco tempo che purtroppo ci è rimasto per vincere una sfida importante, la sfida dei cambiamenti climatici. E non siamo solo noi a dirlo: i cambiamenti climatici sono la sfida principale della strategia *green new deal* tutte le politiche afferenti a questo obiettivo primario ora fanno parte e afferiscono al Mite. Mi riferisco alla politica delle emissioni, e quindi alla qualità della nostra aria, allo sviluppo sostenibile, alla mobilità *green*, alle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, senza dimenticare la base più importante e la missione storica del Ministero: la valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, la conservazione delle aree naturali protette e della biodiversità e poi l'economia circolare, le bonifiche, la difesa del territorio e la lotta ai danni ambientali. Per noi del MoVimento 5 Stelle il Mite è il Ministero che pone come centralità la transizione ecologica e solidale, in quella che è ormai l'era della resilienza, e con consapevolezza affronta una sfida non solo ambientale, ma anche soprattutto sociale, confrontandosi con grande apertura e avendo a cuore il futuro delle nostre generazioni. In questi mesi abbiamo visto che è stato firmato l'atto sull'obiettivo della direttiva 2021, che dà degli indirizzi per la conservazione della biodiversità agli enti parco nazionali e alle aree marine protette. È stato ribadito il concetto di proteggere e ripristinare la biodiversità e assicurare il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare, si fa riferimento agli insetti impollinatori, dai quali dipende oltre il 70 per cento della produzione agricola per la nostra alimentazione. È un grande inizio perché stiamo finalmente quantificando

C'è un'ulteriore notizia degli ultimi giorni: l'inserimento del Parco Nazionale dell'Arcipelago toscano e quello delle Foreste Casentinesi nella *green* *list* dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. natura. È un riconoscimento importante - come ha commentato il ministro Roberto Cingolani - perché fa onore all'Italia, un Paese dalla natura magnifica che sa valorizzare questa preziosissima risorsa. È un riconoscimento non solo in termini di biodiversità, ma anche della gestione complessiva che è stata effettuata e ci incoraggia ad ampliare la rete delle aree protette e dei parchi nazionali italiani, che saranno anche trattati e i protagonisti del Piano nazionale di ripresa resilienza. Barry Commoner, un famosissimo ecologista, diceva sempre che non ci sono pasti gratis in natura. Lui era un ecologista. Ma poi il grandissimo economista Milton Friedman ha parlato del costo opportunità. Il risultato era sempre lo stesso. L'opportunità alla fine significa che, se noi prendiamo un qualcosa, sicuramente sarà la società a rinunciare all'opportunità di destinare le medesime risorse a qualche altro uso. Vogliamo dire

- a un sistema che deve essere ecologico. Perciò parliamo di transizione ecologica.

che abbiamo bisogno di semplificare e utilizzare, ma poi anche di verificare ciò che fanno. Occorre vigilanza perché in questo modo possiamo capire quali sono gli imprenditori veramente virtuosi che hanno fatto per bene le cose e non hanno fatto *greenwashing*. Sono quelli che stanno lavorando per costruire una nuova Italia. *(Applausi)*, e che noi non vogliamo fermare.

Dobbiamo fare questo perché il prezzo di ciò che prendiamo dal pianeta deve essere pagato: tutto ciò che è preso dal sistema ambiente, anche in modalità gratuita, ha un costo.

che gli uomini producono cose inutili e ad alto costo energetico e che non crede siano necessari telefonini sempre più potenti. Al contrario, è necessario sistemare l'ecosistema perché lo abbiamo rovinato. Invecchiare, vivere a lungo va bene se la salute è buona e vivere in tanti sul pianeta significa cercare equilibri sostenibili. «Ecco perché sono orgoglioso - diceva - di appartenere al gruppo di scienziati che fa scienza per quelli che verranno dopo di noi». Egli non è solo uno scienziato, ma anche un Ministro, quindi noi ci fidiamo di lui e di quello che deve fare. Noi del MoVimento 5 Stelle chiediamo al Governo, al Ministro e al nuovo Ministero ci basterebbe che fosse applicato il principio di precauzione. Si tratta di un principio del 1982, inserito nella Carta mondiale della natura. Esso spiega che le attività che comportano un elevato grado di rischio per la natura devono essere precedute da un esame approfondito; i loro promotori devono dimostrare che i benefici derivanti dall'attività prevalgono sui danni eventuali alla natura e, qualora gli effetti nocivi di tali attività siano conosciuti in maniera imperfetta, esse non dovranno essere intraprese. Credo sia chiaro. Dobbiamo, quindi, gestire situazioni di pericolo ambientale, che molto spesso sono sconosciute, complesse e accompagnate da incertezza, a volte anche scientifica, e da un margine di rischio e di errore.

che cambia l'assetto dei suoi Ministeri. Ogni volta che si insedia un Governo, alcuni Ministeri cambiano il proprio assetto interno e questo ovviamente determina disagi, rallentamenti e problemi per tutto il sistema istituzionale, per la gestione degli affari correnti e per tutto quello che di straordinario, purtroppo anche in funzione del Piano nazionale di ripresa si deve comunque portare avanti con efficacia ed efficienza. Curioso che i Ministeri che vengono modificati nella loro nomenclatura e costituzione siano i due Ministeri che si occupano di beni comuni: quello che si occupava, si occupa e si dovrebbe occupare di tutela del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese e quello che si deve occupare di tutela dell'ambiente. Questi due Ministeri, che rappresentavano presidi di cittadinanza, perché servivano a custodire in maniera disinteressata il patrimonio dei cittadini, adesso vengono orientati verso

transizione ecologica. Siamo passati dalla tutela dell'ambiente, del territorio e del mare alla tutela di un processo economico e produttivo, contemplato nella transizione ecologica, che dovrebbe abbinare il principio di tutela a quello dell'efficienza e della competitività energetica. Ma come si sposa il concetto di competitività energetica con quello di tutela dell'ambiente? La stessa cosa dicasi per il Ministero per i beni e le attività culturali, che adesso diventa Ministero della cultura, inserendo un coacervo di attività, anche produttive, che sottraggono centralità all'azione di tutela e conservazione del patrimonio. Tutto questo fa parte di un disegno neoliberista

tutelati solo se parte di processi economici, quindi non come valori, identità e priorità assolute per la cittadinanza attiva dei nostri figli e delle generazioni future. L'Alternativa C'è voterà no al provvedimento in esame. Signor Presidente, non condivido l'entusiasmo che ha accompagnato l'impianto di questo super Governo di tutti, soprattutto su quella che è la parte che ha entusiasmato di più e ha convinto il MoVimento 5 Stelle a dare l'appoggio a questo Governo. Mi riferisco alla creazione del cosiddetto Ministero della transizione ecologica.

sovrastrutturato rispetto agli altri Ministeri, a cui avrei sicuramente aggiunto anche quello della salute, di cui dopo vi dirò) ma perché quella che a questo punto mi appare come una scatola che si sovrappone perde la denominazione di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È stato detto anche dalla collega De Petris in maniera molto chiara, anche se lei voterà a favore e io mi troverò a votare contro. Il concetto è lo stesso. Non posso dimenticare che nel 2013 si voleva eliminare il Ministero dell'ambiente e oggi, in un gioco delle tre carte, vedo che il Ministero dell'ambiente è stato eliminato. Questo non può non suscitare in me - e nelle persone che come me voteranno no un'inquietudine, perché nel CITE troviamo tutti gli altri Ministeri che si occupano dell'energia, dell'industria, ma non si occuperanno dell'ambiente. Si dice che le competenze saranno le stesse, ma, come ho detto in fase di illustrazione degli emendamenti, le parole non sono forma, sono sostanza. Le parole concorrono a formare la nostra percezione della realtà, e se oggi ancora diciamo l'ex Ministero dell'ambiente, domani ci saremo dimenticati dell'esistenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A A questo mi oppongo seriamente e strutturalmente, perché ritengo che se qualcuno avesse chiesto di togliere la tutela dell'ambiente dalle prerogative legislative del Governo, dalla Costituzione,

alle vecchie denominazioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della sanità pubblica, perché l'esperienza di questo anno ci ha dimostrato che quella è l'unica direzione che dobbiamo intraprendere. Nel CITE incluso anche il Ministero della salute, perché l'Organizzazione mondiale della sanità si pone due obiettivi: quello, sì, di superare il male, ma anche di puntare al beneficio di tutti, che solo in un ambiente sano si può ottenere. Per questo motivo annuncio il voto contrario.

Signor Presidente, colleghi senatori, l'ondata di gelo ha devastato nelle notti del 7 e 8 aprile scorso in modo irrecuperabile molte delle coltivazioni agricole nel settore ortofrutticolo e anche cerealicolo del nostro Paese. Pur essendo ancora in corso la raccolta dati, le prime stime indicano che si sono persi raccolti di kiwi, di albicocche, di susine, di pesco, di nettarine, mirtilli, piccoli frutti, nocciole, con timore anche per grano, mais, coltivazioni orticole, pascoli, la produzione del foraggio maggengo, con un'incidenza di danni che va dal 40 al 60-70 per cento della possibile produzione. È indispensabile che il Governo dichiari da subito lo stato di emergenza ed assegni risorse certe, al fine di sostenere gli agricoltori colpiti da questa imprevedibile e gravissima calamità naturale. Occorre poi far accedere immediatamente tutte le aziende agricole colpite al Fondo di solidarietà nazionale,

ferma restando la necessità di un intervento strutturale su questo argomento che è fondamentale. Presidente, sappiamo tutti che le compagnie di assicurazione non sono certamente degli enti di beneficenza e, quindi, con il crescendo degli eventi da indennizzare, le tariffe sono costantemente in aumento e le condizioni di polizza sono sempre peggiorative per gli agricoltori e per i contadini. Per far questo occorre, fin da subito, incrementare i fondi per la gestione del rischio per il biennio 2021-2022, utilizzando eventualmente le prossime misure sullo scostamento che andiamo ad approvare proprio in questi giorni. Dico anche che a volte copiare bene è istruttivo e significa anche guardarsi attorno. La vicina Francia sul tema gelate nei giorni scorsi ha già istituito un Fondo di solidarietà eccezionale da un miliardo di euro e assegna una busta emergenza entro quindici giorni ai prefetti per fornire supporto immediato alle aziende agricole in difficoltà. Vorrei anche ricordare i 150.000 lavoratori agricoli, stimati dalle associazioni sindacali, che rimarranno senza lavoro a causa delle gelate. Suggeriamo immediatamente un paio di soluzioni:

la seconda è una modifica immediata, come da emendamento che la Lega ha presentato al decreto-legge sostegni, per quanto riguarda la legge n. 223 del 1991, in modo tale che ci sia la possibilità di dare una tutela forte a questi lavoratori in difficoltà. Bisogna decidere subito e in fretta perché è fondamentale intervenire. Non possiamo lasciare gli agricoltori italiani soli in un momento così grave e difficile *(Applausi)*.

Imperi, nazioni, nazionalismi, ragion di Stato, ipocrisia, potere sono gli altari su cui si immola la propria umanità, spargendo il sangue degli innocenti sepolti nelle pieghe oscure della storia, in modo da cancellarne per sempre il ricordo e poter girare lo sguardo altrove ancora una volta. Signor

davanti a noi, impietosamente quelle vittime ci guardano negli occhi e ci illuminano in questa centoseiesima ricorrenza del genocidio e dei precedenti crimini commessi contro gli armeni. Il 24 aprile è il giorno del ricordo dell'inumana crudeltà subita da inermi uomini, donne e bambini. Oggi, domani e nei giorni futuri non dimenticheremo chi ha gettato la sua anima agli inferi: l'allora impero ottomano e i suoi alleati. Tale crimine ha mostrato come sterminare scientificamente l'uomo, così avvenne poi per la Shoah e per agli altri crimini contro l'umanità. siamo vicini al popolo armeno, con il nostro cuore afflitto, con la nostra anima dolente, ma con la determinazione affinché tutti sappiano e mai nessuno più pratichi e concepisca tali efferati, disumani crimini contro l'umanità, per la pace e il rispetto di noi stessi.